n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport»

Senatori, con profonda emozione desidero oggi rivolgere un commosso pensiero a Diana De Feo. Una vera amica, oltre che una stimata collega, che tutti noi ricordiamo tra gli scranni di questa Assemblea nella XVI legislatura. Donna brillante, di vivace intelligenza e profonda cultura, Diana De Feo ha sempre inteso il giornalismo e l'impegno culturale come una missione di vita. Passioni ereditate dal padre Italo, storico capo dell'ufficio stampa del Comitato di liberazione nazionale, che Diana ha saputo interpretare con garbo, professionalità e costante dedizione. Dalla ventennale collaborazione con l'«Almanacco del giorno dopo» ai tanti servizi realizzati come inviata speciale del TG1 per l'arte e la cultura, il suo è sempre stato un giornalismo accurato, di qualità, una professione vissuta in ogni occasione con rigore, serietà e onestà intellettuale, espressione di un amore incondizionato per la ricerca e la narrazione della verità. Quella stessa prospettiva di valori ha contraddistinto il suo impegno politico e l'attività parlamentare di senatrice. Ho ancora chiaro il ricordo del suo appassionato impegno come relatrice del disegno di legge, approvato poi all'unanimità da questa Assemblea, sulla non sequestrabilità dei beni artistici prestati all'Italia per l'esposizione al pubblico da Stati o da altri soggetti stranieri; un provvedimento che all'epoca non ha potuto completare il suo *iter*, ma che nelle legislature successive è stato oggetto di analoghe iniziative da parte di quasi tutti gli schieramenti politici. La difesa del nostro patrimonio artistico, in Italia e all'estero, è stata una costante del suo impegno pubblico, anche dopo essersi ritirata dalla politica attiva. Tante sono le iniziative culturali legate alla preservazione e alla promozione delle ricchezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche della Campania e di Napoli, in particolare, che l'hanno vista protagonista. Proprio Napoli, la città che l'aveva adottata, era diventata parte integrante dell'identità di Diana; aveva contribuito a plasmare quella spontaneità e quella energia vitale e contagiosa che tutti noi amavamo in lei. La notizia della sua improvvisa scomparsa è stata motivo di profondo dolore per tutti coloro che, come me, hanno avuto il privilegio di conoscerla, di lavorare al suo fianco e di lasciarsi conquistare dalla sua passione e autenticità. Con Diana De Feo ci lascia una donna di grande umanità, sempre aperta al dialogo e alla condivisione delle idee. Una personalità sincera, spontanea, libera; un'amica che ho sempre ammirato per coerenza di pensiero, generosità e forza di carattere. In ricordo della senatrice Diana De Feo, invito pertanto l'Assemblea a stringersi al dolore del marito Emilio Fede, delle figlie Sveva e Simona, dei nipoti e delle persone a lei care e ad osservare un minuto di silenzio.

L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro della difesa sulla conclusione della missione militare italiana in Afghanistan». Ha facoltà di parlare il ministro della difesa, onorevole Guerini. Signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, desidero, in primo luogo, ringraziare questa Assemblea per l'opportunità di poter illustrare, mentre è in corso il completamento del rientro in patria del nostro contingente, le circostanze che ci hanno portato alla conclusione della missione in Afghanistan, il più importante impegno militare delle nostre Forze armate fuori dai confini nazionali dalla Seconda guerra mondiale. Lo scorso 8 giugno mi sono recato ad Herat per l'ultimo ammaina bandiera del nostro contingente: un momento toccante e straordinario con cui si è chiuso un capitolo significativo della nostra storia. Oggi le nostre Forze armate sono ormai prossime alla conclusione di un imponente sforzo logistico ed operativo, condotto con puntualità e sicurezza: un'altra eccezionale dimostrazione di professionalità da parte dei nostri militari, ai quali va il più sentito ringraziamento, mio e del Governo, per la serietà e l'efficacia con cui quotidianamente svolgono il proprio ruolo per la sicurezza, sia nei teatri operativi che sul territorio nazionale. Non è semplice condensare vent'anni di sforzo nazionale in alcune decine di minuti di intervento, così come è parimenti arduo dare la meritata visibilità alla dedizione e allo spirito di sacrificio che hanno animato l'agire dei nostri oltre 50.000 uomini e donne in uniforme che si sono avvicendati in questi lunghi anni, affiancati dal personale del Ministero degli affari esteri e di molte organizzazioni non governative, e che hanno contribuito a dare il massimo lustro al nostro Paese. Di fronte a voi e certo di interpretare i vostri sentimenti, voglio ricordare con gratitudine i 723 feriti e con profonda commozione le 53 vittime italiane che hanno perso la vita al servizio della Repubblica per portare stabilizzazione e pace in Afghanistan.

L'estremo sacrificio di chi oggi non è più tra noi non deve essere vano e sarà alla base delle iniziative che continueremo a portare avanti per non disperdere i risultati ottenuti. Il loro ricordo sarà indelebile, certamente nel cuore delle loro famiglie, cui va il mio pensiero più affettuoso, ma anche, ne sono certo, per l'intera comunità nazionale. La decisione sulla conclusione della missione *Resolute Support* è stata assunta dal Consiglio atlantico, come largamente pubblicizzato, lo scorso 15 aprile, su proposta di Washington, in applicazione degli accordi tra l'amministrazione americana e il movimento talebano sottoscritti a Doha nel febbraio del 2020. È stata una decisione non facile, arrivata al termine di un di un periodo di profonda riflessione nell'ambito dall'Alleanza sul futuro della missione. Durante tale periodo, ho spesso ribadito, nell'ambito delle riunioni ministeriali, la necessità di essere aderenti al principio *"in together, adjust together, out together"*: siamo arrivati insieme, ci siamo adattati insieme, concludiamo insieme. Un principio che ha caratterizzato l'intera permanenza della NATO in Afghanistan. Abbiamo perciò avviato il rientro dal Paese asiatico, dove le forze alleate operavano fin dal 2001, all'indomani dell'11 settembre, quando l'attacco terroristico alle Torri gemelle sconvolse il mondo, cambiando radicalmente il paradigma della sicurezza collettiva. Non è un caso che ciascuno di noi ricordi esattamente dov'era e cosa stava facendo quel giorno, sentendo chiara la percezione che il mondo non sarebbe stato più come prima. Gli Stati Uniti invocarono, per la prima volta nella storia della NATO, l'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico, chiamando gli alleati ad un'assunzione di responsabilità, a cui l'Italia non si sottrasse, confermando la scelta di essere produttore di sicurezza e non solo fruitore e risultando, a seguito di una decisione condivisa dal Parlamento, tra i primi Paesi a fornire un contributo concreto nella lotta al terrorismo globale. Per dare la giusta collocazione ad un impegno durato un ventennio, occorre ricordare che lo sforzo della comunità internazionale non si è concretizzato unicamente in un susseguirsi di attività militari, di cui l'operazione Resolute support ha rappresentato l'ultimo capitolo. In questi venti anni, infatti, l'intervento in Afghanistan è stato essenziale per la ricostruzione del tessuto democratico e istituzionale del Paese, che dal 2004 ha una nuova Costituzione, e per ripristinare e rafforzare quei diritti civili che il regime talebano aveva violentemente soppresso, in particolare nei confronti delle donne. La dimensione militare, particolarmente estesa e per certi versi prevalente in termini di narrazione, è stata comunque una delle direttrici fondamentali dello sforzo internazionale, in particolare, soprattutto negli ultimi anni, per la costruzione in Afghanistan di un apparato di sicurezza nazionale in grado di garantire la stabilità e il controllo del territorio. Si tratta di attività che hanno visto l'Italia ricoprire un ruolo da protagonista. altro settore fondamentale, a cui la componente militare ha garantito l'essenziale cornice di sicurezza, ha visto profondere oltre 76 miliardi di dollari di aiuti internazionali in attività di *state building*, con l'obiettivo di garantire lo sviluppo economico e la disponibilità di servizi a favore della popolazione. Il coinvolgimento del nostro Paese nelle operazioni militari volte alla stabilizzazione dell'Afghanistan è iniziato il 7 ottobre 2001. Con l'avvio da parte degli Stati Uniti dell'operazione Enduring freedom iniziava infatti un impegno, che ci ha visto significativamente presenti, in piena coerenza con il sostanziale, generoso e solidale contributo, che l'Italia da sempre garantisce a favore della sicurezza internazionale. Nel 2005 la missione ISAF, che subentrò ad Enduring freedom, affidò all'Italia il ruolo di *lead nation* nella provincia occidentale del Paese, nel quadro dell'espansione della missione. Ciò includeva anche la responsabilità di farsi carico della gestione del *provincial reconstruction team* (PRT), ubicato ad Herat. definitivamente conclusasi nel 2014, ha messo in luce la proficua cooperazione tra la componente civile del Ministero degli affari esteri e della cooperazione Tale sinergia ha permesso, in nove lunghi anni, di realizzare un numero considerevole di interventi, di cui ha beneficiato la popolazione afghana, soprattutto quella delle zone più rurali del Paese. Giusto per dare una connotazione concreta a questo impegno, ritengo doveroso evidenziare che, durante il periodo in cui l'Italia ha avuto la responsabilità della provincia di Herat, il nostro personale ha portato a termine progetti di cooperazione civile e militare, per un corrispettivo di oltre 46 milioni di euro, che hanno incluso la costruzione di 82 scuole, 37 strutture medico-ospedaliere, 784 pozzi e la realizzazione di più di 100 chilometri di strade e di oltre 30 infrastrutture per le forze di sicurezza e le varie istituzioni afghane. tutte opere rilevanti, che rappresentano un risultato, che testimonia appieno e conferma ulteriormente gli importanti obiettivi conseguiti dal nostro Paese in Afghanistan, soprattutto nel fornire risposte concrete agli effettivi bisogni della popolazione, adottando sempre il riconoscimento e la promozione delle priorità di quelle comunità. Sono insegnamenti di cui abbiamo fatto tesoro e che oggi contraddistinguono il nostro operare coeso in tante aree di crisi, dove la Difesa è fortemente impegnata, come ad esempio l'Iraq o il Sahel. Dal primo gennaio 2015, la NATO ha lanciato la missione Resolute support, che si avvia appunto alla conclusione. È un'operazione non-combat, incentrata sull'addestramento, la consulenza e l'assistenza alle forze di sicurezza afghane. La cornice giuridica della missione venne fornita dallo Status of forces agreement (SOFA), firmato a Kabul il 30 settembre 2014 e successivamente ratificato dal parlamento afghano il 27 novembre dello stesso anno. Questo accordo definì, in piena intesa con le istituzioni afghane, i limiti, i termini e le condizioni entro i quali le forze NATO erano autorizzate a operare nel Paese, così come il mandato della missione e le attività da compiere. La consistenza numerica delle truppe dispiegate in Afghanistan nell'ambito di questa missione si è attestata complessivamente attorno alle 9.600 unità, cui l'Italia ha contribuito con la presenza qualificata di oltre 900 militari e la responsabilità della provincia di Herat. Nel corso dell'ultimo quinquennio i contingenti nazionali alternatisi in Afghanistan hanno condotto attività di addestramento, consulenza e assistenza a favore della controparte afghana in molti settori; oltre a quello prettamente operativo, anche in ambiti complementari, come ad esempio la pianificazione finanziaria e la logistica. Complessivamente sono state condotte oltre 53.000 attività (un numero che credo non necessiti di commenti), tutte di elevatissimo livello, con l'addestramento diretto o indiretto di più di 20.000 militari afghani. Rileva infine, relativamente al mandato del nostro contingente, la continuazione delle attività nella sfera della cooperazione civile e militare, volta al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione; impegno che si è tradotto in 2.200 progetti per un valore di 12 milioni di euro, che portano il totale complessivo, dal 2004 a oggi, a circa 58 milioni di fondi nazionali impiegati a favore delle comunità afghane. Tornando ora alla decisione presa a Bruxelles nell'aprile scorso, come ho detto, non è stata certo facile. L'Alleanza aveva ben chiaro che restare ci avrebbe quasi certamente portati a un ritorno del confronto militare con i talebani, che già si predisponevano a un'ampia offensiva di primavera, di fatto portando a un deterioramento delle condizioni di sicurezza e snaturando la missione Resolute support, dimensionata sugli obiettivi che erano stati condivisi con le istituzioni afghane, cioè addestramento e consulenza. Questo è alla base delle decisioni dell'Alleanza, in linea peraltro con le aspettative degli accordi di Doha che ho citato in precedenza, proprio per ridurre il rischio, comunque presente, di un aumento della violenza e ben consapevoli delle problematiche associate a un'attività di rientro. Voglio condividere con voi la considerazione di quanto sia infatti complessa, in termini organizzativi e di pianificazione, anche un'attività di ripiegamento come quella che stiamo conducendo, forse ancor più dello stesso avvio di una missione. È proprio per questo che oggi il mio impegno come Ministro della difesa è volto innanzitutto a effettuare, di concerto con gli alleati, il rientro ordinato e sicuro del nostro contingente in patria. Posso affermare che le operazioni stanno procedendo, dal punto di vista militare, secondo i piani stabiliti, con il rientro del personale e l'afflusso dei materiali dall'Afghanistan verso i poli logistici (porti e aeroporti) in vari Paesi della regione, per il successivo caricamento su vettori navali e aerei che effettueranno le loro tratte di ritorno verso l'Italia. A oggi sono stati rimpatriati 280 nostri militari e sono già defluiti dal teatro operativo afghano più del 70 per cento dei mezzi e dei materiali verso l'Italia. In questo contesto, in coordinamento con i comandi afghani, è stata valutata anche l'opportunità di lasciare a disposizione delle forze armate e di sicurezza locali parte delle sistemazioni logistiche e dei materiali ritenuti utili da parte loro. Uno sforzo significativo, che il Comando operativo di vertice interforze (COI) difesa ha orchestrato e sta conducendo efficacemente e che si concluderà a breve secondo la pianificazione. Oltre a essere impegnata nel rientro del contingente nazionale, la Difesa sta facendosi carico parallelamente anche di un'attività di trasporto umanitario del personale civile afghano che ha collaborato con le forze italiane, denominata "Operazione Aquila". I nostri collaboratori, al termine delle operazioni di arrivo, accoglienza e profilassi medica, con lo svolgimento della quarantena presso strutture civili e militari, saranno inseriti nel sistema di accoglienza e integrazione nazionale, a cura del Ministero degli interni. A oggi, il personale afghano che ne ha fatto richiesta e che si è dimostrato in possesso di tutti i requisiti consta di 228 tra collaboratori delle Forze armate e loro familiari, di cui 224 sono già in Italia. La definirei un'impresa nell'impresa che ben rappresenta, ancora una volta, la nostra vicinanza e la nostra realtà nei confronti del popolo afgano, uno sforzo doveroso per tutelare l'incolumità dei tanti cittadini afgani che negli anni hanno assistito a vari livelli il nostro personale e che sono stati determinanti per la realizzazione dei risultati che ho precedentemente elencato. È questo un chiaro messaggio: chi lavora con l'Italia non viene abbandonato. Mentre procedono le operazioni di conclusione della missione, ci siamo posti insieme agli alleati anche l'obiettivo di continuare a supportare le istituzioni repubblicane e il popolo afgano nelle forme e nelle modalità che saranno definite sia in ambito NATO che in una possibile dimensione bilaterale. La recrudescenza di violenza, come vi anticipavo, era prevedibile e, in parte, aspettata, ma sembra essere principalmente diretta a esercitare pressione sulle forze di sicurezza afgane in vista della ripresa dei colloqui di pace. Ciò non significa che l'attuale situazione sul terreno non sia per noi, così come per tutti gli alleati, fonte di preoccupazione. Il livello della violenza è aumentato e gli attacchi delle componenti militari e oltranziste del movimento talebano hanno come loro obiettivi non solo, come detto, le forze di sicurezza afgane e il controllo di alcune province, ma anche esponenti della società civile. Non meno rilevante, inoltre, è la minaccia posta dal terrorismo jihadista e dalle sue diramazioni nel Paese, su tutte Isis-Khorasan, che continua ad avere una forte capacità di richiamo sulle province più povere che in maniera insidiosa hanno ripreso a condurre attività cinetiche. In questo complesso contesto le istituzioni repubblicane dell'Afghanistan sono chiamate oggi a tutelare la democrazia e assicurare la tenuta stessa del Paese; le istituzioni che certamente hanno beneficiato del supporto internazionale, che ne ha garantito una maggiore solidità. Tale sfida delicata, in ogni caso, come avvenuto negli ultimi venti anni, sebbene con modalità diverse, vedrà la NATO e gli altri *partner* internazionali impegnati a supporto delle forze di sicurezza afgane, cui sarà assicurato *in primis* il sostentamento economico e finanziario. Ci si potrebbe chiedere in che forma l'Alleanza intenda proseguire il suo sforzo. È una domanda legittima a fronte dell'impegno profuso fino ad oggi e dei sacrifici che anche il nostro Paese ha sostenuto in questo contesto con un ruolo sicuramente da protagonista. Nel corso della riunione ministeriale di esteri e difesa, cui ho partecipato insieme al ministro degli esteri Luigi Di Maio e che ha sancito il termine di Resolute support, le Nazioni hanno deciso che l'obiettivo dell'impegno NATO nel *post* missione è preservare al meglio quanto sinora conseguito, continuando a contribuire allo sviluppo delle istituzioni afgane di sicurezza e difesa, affinché il Paese non diventi nuovamente un paradiso sicuro per il terrorismo. Ciò serve anche a contrastare la narrazione dell'abbandono, che darebbe unicamente forza alle posizioni estremiste. Il nuovo concetto di supporto da parte della NATO prevede tre componenti: la costituzione dell'ufficio dell'Alto rappresentante civile della NATO, incarico ricoperto oggi da un nostro connazionale, l'ambasciatore Pontecorvo; il sostegno alla funzionalità dell'ospedale e dell'aeroporto di Kabul, la cui sicurezza è prerequisito essenziale per mantenere la presenza della componente diplomatica; la formazione, intesa come addestramento e sviluppo capacitivo, fuori dal Paese delle forze afgane di difesa e di sicurezza, con particolare attenzione alle forze speciali, che si sono dimostrate fondamentali per il contrasto ai talebani e alle formazioni terroristiche. Ad oggi l'Alleanza, come da comunicato finale del recente *summit* della NATO, ha confermato di fatto la volontà di mantenere un impegno significativo anche attraverso l'alimentazione del *trust fund* destinato a supportare le forze di sicurezza afgane, al momento fino al 2024. Siamo, perciò, in una fase nuova in cui tutti gli alleati, anche se con diverse sfumature, stanno dando segnali convergenti circa la volontà di proseguire il loro impegno con modalità coerenti con il nuovo scenario. La Difesa italiana, insieme agli altri Dicasteri interessati, sta partecipando attivamente alle interlocuzioni in atto, allo scopo di individuare le forme migliori per un nostro ruolo attivo nel futuro impegno dell'Alleanza, capitalizzando la credibilità ottenuta in questi vent'anni. Aggiungo, inoltre, che, nel corso dei miei frequenti contatti con i colleghi Ministri della difesa, sto verificando le rispettive posizioni nazionali per individuare possibili sinergie, soprattutto per quanto riguarda la formazione fuori dal Paese delle forze afgane. Nel frattempo stiamo finalizzando l'accordo quadro con il Ministero della Difesa di Kabul, che si pone come strumento abilitante e quale imprescindibile base giuridica per avviare future attività sul piano bilaterale. Non lasceremo di conseguenza alcuna progettualità intentata per non disperdere i risultati ottenuti in quattro lustri di gravoso impegno, sia sul piano della sicurezza e dello sviluppo delle forze locali che nel campo dei diritti umani, della parità di genere e delle libertà civili. Tuttavia, oggi, a fronte della cessazione della presenza militare internazionale nel Paese, è necessario che il *focus* dell'azione dei Paesi *framework* NATO che hanno assunto le maggiori responsabilità dello sforzo alleato continui sul piano politico diplomatico e della cooperazione civile, con l'intensità e la continuità necessarie per sostenere il governo repubblicano e la popolazione afghana. Per questo fine ritengo che la presenza delle rappresentanze diplomatiche internazionali nel Paese sia essenziale nello scenario *post* anche per segnalare alle frange più radicali del Movimento talebano che la comunità internazionale non intende accettare passivamente che le lancette dell'orologio vengano riportate indietro di un ventennio. In questo senso non verrà a mancare il supporto del Ministero della Difesa per la tutela del personale diplomatico e della nostra rappresentanza, come pure sarà valutato il possibile coinvolgimento per corroborare l'architettura di sicurezza della capitale. Ho voluto evidenziare gli elementi di criticità con cui la comunità internazionale e l'Afghanistan si devono confrontare, ma devo anche sottolineare alcuni elementi di significativa positività. Mi riferisco innanzitutto alle forze afgane che dopo l'iniziale e comprensibile senso di smarrimento sembrano ora avere interiorizzato la necessità di prendere in mano la loro sicurezza e di essere in grado di reggere l'urto. Esse sono il risultato concreto del nostro sforzo, in particolare con il Resolute support,il cui scopo era proprio quello di favorire una crescita di competenza e autonomia nei colleghi delle Forze armate e di sicurezza afgane. Si tratta oggi di 186.000 militari e di 121.000 appartenenti alle forze di sicurezza del Ministero dell'interno che sono stati in larga parte addestrati ed equipaggiati dalle forze NATO e che già in questi momenti stanno mettendo a frutto efficacemente ciò che hanno appreso. Questo è sicuramente un risultato della nostra presenza in quel Paese, così come sono risultati concreti tutti i passi avanti fatti dal punto di vista sociale, in particolare per quanto riguarda i diritti civili, tra tutti quello all'istruzione, e i diritti delle donne che hanno acquisito ruoli rilevanti nella società afgana. Proprio ieri, nell'ambito di un convegno sulla parità di genere nelle operazioni militari organizzate dal nostro comando operativo interforze, ho avuto modo di incontrare Maria Bashir, procuratore generale della Provincia di Herat, una donna preparata, coraggiosa ed autorevole che come tutte le donne del Paese nel periodo del governo afgano era stata costretta a lasciare il suo lavoro e a rinchiudersi in casa. Oggi, con coraggio e non senza rischi, svolge questo importantissimo ruolo nella società afgana. Questo mi porta a chiedermi e a chiederci cosa sarebbe stato l'Afghanistan senza questi venti anni di presenza e di lavoro fianco a fianco con i governanti e la popolazione e quale sarebbe stato l'impatto sul quadro di sicurezza internazionale. Il nostro lavoro è stato importante per quel Paese, per la sua popolazione e anche per la nostra sicurezza. La decisione di concludere la missione non è un abbandono del campo; le missioni iniziano, si sviluppano, si adattano al mutamento degli scenari - e l'Afghanistan ne è una plastica dimostrazione - si concludono o meglio, come in questo caso, evolvono individuando forme diverse di supporto. È però essenziale che l'impegno della comunità internazionale e del suo *focus* sull'Afghanistan non vengano mai meno e oggi in particolare si concentrino sulla necessità di riprendere e rafforzare i negoziati di pace intraafgani. Infatti la soluzione del conflitto, assieme alla continuazione del supporto alle forze di sicurezza, è la via principale per un Paese realmente pacificato, che possa contare sulla stabilità delle sue istituzioni. Ciò detto, mi preme ribadire che oggi il principale impegno, mio e di tutte le articolazioni del Dicastero, è quello del rientro in piena sicurezza del nostro personale in un contesto particolarmente complesso e non privo di rischi. Nell'avviarmi alla conclusione di questo intervento, ritengo doveroso evidenziare che le Forze armate, dopo questi vent'anni, sono professionalmente cresciute, grazie alle esperienze svolte in un contesto di elevata complessità come quello afgano: abbiamo migliorato le capacità di proiezione, di comando e controllo, la preparazione professionale e gli equipaggiamenti di mezzi, nel confronto con un ambiente operativo estremamente sfidante. I militari italiani hanno operato con successo, bilanciando la nostra propensione alla vicinanza alla popolazione locale con la capacità di condurre, al fianco delle forze di sicurezza afgane, operazioni militari ad alta intensità. un lascito importante, che le Forze armate sono state in grado di capitalizzare e di reimpiegare in maniera estremamente efficace, in tutte le circostanze operative che le vedono impegnate oggi nei numerosi teatri di crisi in cui l'Italia svolge un'apprezzata opera al servizio della sicurezza e della stabilità internazionale. Permettetemi in conclusione, anche per questo, di esprimere ancora una volta la gratitudine delle nostre istituzioni nei confronti dei nostri militari, delle nostre donne e dei nostri uomini in uniforme *(Applausi)*, per il prezioso lavoro che fanno e per come lo fanno. Dovunque siano impegnati nel mondo a tutela della sicurezza internazionale, dimostrano costantemente, come avvenuto nei vent'anni della nostra presenza in Afghanistan, di credere profondamente nel loro lavoro per contribuire, anche a costo di importanti sacrifici, alla realizzazione di condizioni di vita migliori nelle terre in cui operano, luoghi che spesso purtroppo hanno visto tanta sofferenza. L'Italia intera dev'essere loro grata, perché tramite loro il Paese ha dimostrato (e continua a farlo) di essere sempre all'altezza delle sfide che siamo chiamati a fronteggiare. *(Applausi)*.

(affascinanti e terribili, per altro verso) nel 2005, quando quel Paese ci emozionò per la prima volta con il voto elettorale e la partecipazione femminile. Ricordo molte di quelle coraggiose, ma questo è il passato. Questa missione è una delle più lunghe (per gli Stati Uniti è più lunga della guerra del Vietnam), quindi è chiaro che le preoccupazioni che le preoccupazioni sono molte: per esempio, il cessate il fuoco negoziato tra americani e talebani copre solo le forze internazionali, quindi va esteso. Inoltre, mentre gli attacchi alle forze internazionali sono diminuiti, la violenza interna contro la popolazione civile è di molto aumentata. molto aumentata. Talebani moderati non ne conosco, però può darsi che si siano moderati nel corso degli anni. Pertanto, da questo punto di vista, la preoccupazione di tornare indietro su temi fondamentali come i diritti umani (per tutti, non solo per le donne) è palpabile, così come la violenza che esplode sempre di più, rivendicata da strani gruppi islamici non moderati (non so come li vogliamo chiamare).

Noi però non possiamo abbandonare questo terreno. Una delle proposte che le donne e parte della società civile hanno fatto al Parlamento europeo è l'istituzione di una commissione internazionale di inchiesta, analoga ad altre che ci sono in varie parti del mondo, per avere qualche testimone che rimanga sul terreno a difesa di quello che è stato conquistato fin qui e che non dovrebbe essere cancellato con un ritorno barbarico. le faccio due proposte. La prima, quella della commissione, nel Consiglio dei diritti umani di Ginevra, che si è aperto pochi giorni fa e che si chiuderà il 15 luglio, ha già ottenuto il sostegno di altri Paesi.

che la Norvegia si è impegnata a portare al Consiglio di sicurezza, di cui è membro. Sono gli ultimi sei mesi di presenza italiana nel Consiglio dei diritti umani e per gli afgani e noi stessi credo sarebbe utile e un buon passaggio che questa iniziativa prendesse piede, sospinta dal Governo italiano (insieme agli altri, evidentemente), per non sembrare quelli che fanno le valigie e vanno via. Che

Soprattutto, come capita ogni tanto, mi sono chiesto: vale la pena che dica quel che penso o debbo cercare di avere l'ipocrisia che a volte noi politici abbiamo? (Sto parlando di me, riferendomi politici). A questo punto, per quanto mi riguarda, tanto vale che dica quel che penso: non devo più far carriera, per cui il problema non riguarda le mie prospettive, ma me stesso e quello che penso del futuro del nostro Paese.

senza rendersi conto di come si sta al Governo. Lei, signor Ministro, ha detto le cose che un uomo di Stato deve dire su questo. Noi, che siamo il Parlamento, possiamo dire le cose che condividiamo al cento per cento e anche la realtà delle convinzioni che invece ci mancano. una cosa su cui credo nessun italiano possa discostarsi di un millimetro da quello che ha detto è che le Forze armate italiane hanno dato una prova straordinaria di cosa significa portare il Tricolore in giro per il mondo; lo hanno fatto con azioni militari e di pacificazione, con i Governi di destra, di sinistra o di centro: l'hanno fatto sempre. In questi vent'anni le Forze armate italiane - lei ha fatto bene a ricordarlo - sono cresciute in termini di professionalità, di considerazione e di rispetto nel mondo. E se l'Italia ha ancora un barlume di politica estera, questo è possibile anche e in gran parte per le azioni dei nostri militari nelle missioni di pace.

che si sono sacrificati per la più grande missione fatta da noi come Forze armate italiane dopo la seconda guerra mondiale; è una cosa immensa. Se aggiungiamo a questi caduti quelli di Nassirya e delle altre missioni militari di pace, ci rendiamo conto del prezzo enorme che tante famiglie italiane hanno pagato. Siamo orgogliosi

una risposta al senso della storia. Credo che in effetti questi caduti non siano morti invano, perché ha avuto un senso il percorso che abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto perché, quando si sta in una comunità internazionale, si sta assieme agli altri a combattere per dei principi e per dei valori. Ha avuto un senso, come ricordava la senatrice Bonino dall'alto della sua esperienza e come lei ha detto, che donne che erano emarginate e chiuse in casa siano diventate protagoniste del Parlamento e del Governo del Paese. Ha un senso che i diritti delle persone si siano potuti affermare, ma a questo punto mi fermo qui.

sui diritti delle donne si sono fatti giganteschi passi indietro, che l'esercito afghano - come temo - non sia affatto in grado di stabilizzare sul terreno la situazione e di garantire la sicurezza,

arrestati tutti i candidati presidenziali antagonisti di Ortega. Qualcuno mi ha detto che è una cosa irrilevante: certo, si fanno le elezioni e tutti quelli che si presentano contro di me li faccio arrestare. Abbiamo

buttati in carcere e si perde la chiave, ma tutto questo è irrilevante, perché siamo per i diritti umani. Ho sempre contestato l'idea che possiamo esportare la democrazia come modello:

dire naturali, che i Paesi devono rispettare. Mi rendo conto che la mia è l'espressione di una preoccupazione, alla quale un uomo di Governo non può che rispondere dicendo che queste sono riflessioni che evidentemente si faranno. Temo, tuttavia, che anche l'amministrazione americana, che nasce all'insegna della riscoperta giusta del multilateralismo e del concetto di un Occidente che deve difendere la democrazia, rischia poi, quando certe cose si materializzano, di trovare una strada irta di ostacoli. In ogni caso, signor Ministro, aderisco alla sua impostazione, nel senso che il Governo italiano si è mosso in modo ineccepibile e non poteva fare diversamente: nel momento in cui

lo continuiamo a fare in tante parti del mondo. Dobbiamo anche far capire all'opinione pubblica quello che è importante oggi, per i valori condivisi di cui l'Italia è certamente portabandiera nel mondo.

salutiamo il ritorno a casa dei nostri ragazzi, delle donne e degli uomini delle nostre Forze armate impegnati in Afghanistan dall'ottobre del lontano 2001. A tutti loro va un ringraziamento sentito e caloroso. Profonda vicinanza va, in primo luogo, ai familiari di quei 53 militari che purtroppo, nel corso di quegli anni in Afghanistan, sono rimasti vittime di un attentato o un incidente, in questi giorni non possono che provare un rinnovato profondo dolore nel ricordo dei loro cari che non possono beneficiare del ritiro in corso. Il nostro ringraziamento più sentito va anche a tutte le donne e agli uomini che hanno servito con devozione il nostro Paese e lavorato per la pace e la stabilizzazione di una regione impervia, difficile e pericolosa come l'Afghanistan. Condividiamo il loro sollievo e quello che provano i loro cari a vederli tornare a casa sani e salvi. Attualmente sono 900 i militari che compongono la nostra missione italiana, ma in tutti questi anni sono stati oltre 50.000 i soldati che hanno partecipato all'operazione. Abbiamo passato oltre vent'anni lì, dentro la base militare che è stata il centro delle attività del contingente italiano inviato a suo tempo a causa dell'attentato alle Torri Gemelle, con l'obiettivo di debellare la cellula terroristica di Al Qaida, sconfiggere i talebani e assicurare al Paese il ripristino delle libertà politiche e civili e il normale esercizio dei diritti fondamentali. Ministro Guerini, a vent'anni di distanza è stata una grande emozione veder ammainare il nostro tricolore alla base di Herat. Attraverso quel gesto simbolico è come se avessimo ripercorso velocemente le immagini delle tante azioni pregevoli condotte in questi due decenni dai nostri militari in Afghanistan: il salvataggio di tante vite umane; i numerosi progetti di cooperazione volti a sostenere un popolo afflitto dal terrorismo; i corsi di formazione per giovani e donne; il sostegno alle Istituzioni per spronarle a promuovere processi di democratizzazione; la costruzione di scuole, ospedali, strade e infrastrutture pubbliche, come ha ben ricordato il ministro Guerini nel suo intervento. Tutto questo dopo che per anni il regime dei talebani, in modo del tutto arbitrario, aveva pesantemente segnato il destino del popolo afghano, attraverso una politica reazionaria, basata sull'uso del terrore e della violenza. Ad esempio, aveva inflitto brutali mutilazioni alla popolazione responsabile di piccoli crimini; non aveva esitato a mandare al patibolo persone arrestate per reati di modesta gravità; aveva chiuso le scuole femminili, escludendo le donne dalla vita pubblica; aveva distrutto monumenti archeologici di straordinario valore; aveva vietato musica, film e televisione, obbligando gli uomini a farsi crescere la barba e le donne a usare il *burqa*. Insomma, aveva imposto un fanatismo ideologico basato sull'uso della violenza e della paura. Non c'è da stupirsi se oggi in Afghanistan in tanti guardano con apprensione al ritiro delle truppe internazionali. Molti temono il ripristino di un regime repressivo, oppure lo scoppio di una nuova guerra civile. Purtroppo, i talebani sono ancora forti - lo si vede, ahimè, anche in questi giorni - e lo sono ancora di più da quando l'*ex* presidente Trump ha deciso di trattare il ritiro accordandosi in modo bilaterale soltanto con loro, rafforzandone il potere e indebolendo al contempo il Governo istituzionale afghano, escluso dal tavolo delle trattative. L'accordo bilaterale tra talebani e Washington firmato a Doha nel febbraio 2020 ha messo fine al conflitto tra gli americani e la guerriglia in turbante nero, ma non a quello tra talebani e forze governative. L'accordo per la pace in Afghanistan prevede infatti un ritiro totale dei soldati stranieri, ma non impone un cessate il fuoco, né una riduzione della violenza. Il presidente Biden ha deciso di fare sue le scelte di un progressivo disimpegno degli Stati Uniti in quell'area, voluto e pensato già dal presidente Barack Obama, ma il tutto non è privo di contraddizioni. Infatti, mentre noi occidentali ce ne andiamo, non lasciamo un territorio pacificato. Questo è il motivo per il quale anche noi di Italia Viva siamo preoccupati dalla tempistica del ritiro dall'Afghanistan dei diversi contingenti internazionali. rispettiamo la scelta intrapresa di ritirare le nostre truppe dall'Afghanistan, anche perché siamo consapevoli che viene esercitata nel solco di quell'Alleanza Atlantica che il nostro Paese sta recuperando con l'attuale Governo, dopo una passata fase di ambiguità nei rapporti di politica estera, e vale il principio "*together in, together out*". Allo stesso modo, non possiamo che rilevare i pericoli che si insinuano dietro questa decisione: temiamo che possa essere una partenza prematura e che possa dare il via a una nuova ondata di odio nel Paese. Tutti coloro che hanno aiutato le nostre missioni adesso hanno paura di subire ritorsioni. Il nostro Paese, in modo pregevole, sta già aiutando gli interpreti afghani e, in generale, il personale civile che ha supportato il nostro contingente, provvedendo gradualmente al loro trasporto umanitario. Verranno trasferite in Italia 270 persone, tra collaboratori e relativi familiari, e si sta accertando la possibilità di trasferire ulteriori 400 afghani per il rapporto di collaborazione prestato al nostro contingente negli anni: un intervento nobile, ma naturalmente applicabile soltanto a singoli destinatari. E c'è tutto il resto della popolazione, che ora rischia di pagare le conseguenze della ritirata occidentale, oltretutto in un periodo complicato. Le prime avvisaglie già si sono viste a Jalalabad, nell'Afghanistan orientale, dove uomini armati hanno preso di mira le squadre di vaccinazione, uccidendo diversi membri dello *staff* e ferendone altri tre. L'Italia non dimentica - la cito, signor Ministro - chi in questi anni in Afghanistan ha collaborato con i nostri militari. Ci permettiamo di aggiungere che l'Italia non dimentica neanche l'intero popolo afghano rimaniamo impegnati per la sua pace e la sua salvezza, nonostante la situazione molto complicata. Certo, conforta sapere che la NATO continuerà a fornire formazione e sostegno finanziario alle forze di sicurezza e di difesa nazionali afghane, anche attraverso il mantenimento di rapporti diplomatici, tramite l'ufficio di un Alto rappresentante civile a Kabul, così com'è positiva la previsione di finanziamenti *ad hoc* per garantire il funzionamento dell'aeroporto internazionale in quella tutte previsioni importanti e valide. Adesso bisogna però creare le condizioni affinché il ritiro delle truppe dall'Afghanistan non significhi porre fine ai rapporti con il Paese. È il momento di aprire un capitolo nuovo, confermando l'impegno a rimanere al fianco dell'Afghanistan, del suo popolo e delle sue istituzioni, così da continuare a sostenere il processo di pace in corso e promuovere la sicurezza interna e internazionale, nel tentativo di preservare le conquiste faticosamente ottenute negli ultimi vent'anni ed evitare che il Paese diventi, purtroppo, un serbatoio di possibili futuri attacchi terroristici. Molti afghani - e noi con loro - temono che la pace possa rivelarsi un inganno, con i talebani che non aspettano altro che la partenza degli occidentali per rovesciare un governo fin troppo debole, così da ripristinare il loro regime. Questo non è tollerabile, perché sarebbe una tremenda delusione se un ritiro affrettato aprisse le porte a una nuova epoca oscurantista in Afghanistan. Gli afghani e soprattutto le afghane non se lo meritano e neanche le donne e gli uomini delle nostre Forze armate, che in questi anni tanto impegno e dedizione hanno profuso per la stabilizzazione dell'Afghanistan. *(Applausi)*. Signor Presidente, ringrazio il ministro Guerini per la sua esposizione, che in molti punti mi ha convinto, anche se mi tocca esprimere una critica alla scelta di venire in Aula a cose fatte. Lo so benissimo, non sarebbe cambiato molto: rispondiamo a una logica atlantica e a decisioni cui partecipiamo, ma su cui non possiamo incidere più di tanto. Credo però che questo Parlamento avrebbe meritato di poter svolgere questo dibattito prima dell'avvio del ritiro delle truppe. Non è un fatto formale, ma sostanziale, anche di rispetto verso coloro che hanno tenuto alto il nome e il prestigio non solo delle Forze armate, ma di tutta l'Italia. Mi consenta, quindi, questa critica. Subito dopo voglio invece prendere atto che il mio amico, senatore Casini, ha sentito il bisogno di introdurre il suo ottimo intervento con l'affermazione che doveva dire quello che pensava, quasi che fosse qualcosa che di solito in quest'Aula non si può fare. Siccome concordo con quanto ha detto (voglio ricordare che ha detto che bisogna essere orgogliosi dei nostri soldati, soldati, che sono stati bravi in questi anni di dura missione e che non sono morti invano), c'è bisogno di non avere aspettative politiche, come lei ha detto, presidente Casini, per dire questo? Non è una critica a lei. a lei. Questo è l'aspetto che più mi ha preoccupato in questi anni, cioè il fatto che la nostra missione dovesse essere guardata - da alcuni, non da tutti - con sospetto; - con sospetto; che i nostri soldati e le nostre donne (perché c'erano ragazzi, uomini maturi e donne con le stellette in Afghanistan) non dovessero avere il giusto riconoscimento giorno per giorno da parte dei Ministri della difesa. Vedo la senatrice Pinotti: da lei è stato sempre riconosciuto, come da Guerini, da destra a sinistra; quando si è al al vertice di quella struttura che è il Ministero della difesa ci si rende conto e, al di là delle posizioni politiche, si finisce per apprezzare, difendere e capire lo sforzo e il sacrificio

poter dire apertamente - e fino ad allora non avveniva - che non erano lì solo per costruire strade e distribuire acqua minerale e palloni ai bambini, bambini, ma per una missione di pace che comportava anche il duro combattimento e il rischio della vita. E questo è stato pagato non solo da 53 italiani, italiani, ma anche da 3.600 militari della missione: 53 italiani e 3.600 uomini e donne hanno dato la vita. È giusto È giusto allora interrogarsi: ne è valsa la pena? Me lo chiedo oggi, come me lo sono chiesto quando ero Ministro della difesa. Tutte le volte che mi toccava andare all'aeroporto

È una domanda terribile, che credo ci si sia sempre posti, tutte le volte che ai nostri uomini e alle nostre ragazze e donne con le stellette si chiede di svolgere il loro compito a rischio della loro vita.

più cibo, più licenze, più vantaggi materiali; mi chiesero più elicotteri, per svolgere meglio la loro missione, nella quale credevano e per la quale erano pronti a fare fino in fondo il loro dovere. La risposta me l'hanno data loro, in questa maniera. Quando Quando torna in mente l'opera che hanno svolto in questi anni, non mi sembra che il vantaggio sia stato solo per le donne afghane, per i giovani e gli uomini afghani o per le istituzioni afghane, che si sono giovate grandemente di queste missioni, di questa missione e del sacrificio dei nostri militari. Pensate alle donne, alla donne, alla qualità della vita e al modo di vita prima, durante e - speriamo - dopo, ma anch'io nutro i dubbi che ho sentito aleggiare in quest'Aula. Non è stato solo questo, però: spesso sottovalutiamo l'altro grande risultato, grande risultato, che è di casa nostra, perché quegli uomini e quelle donne che sono andati lì a combattere per la pace

che adesso comanda il rientro in Italia e che ha comandato l'ultima fase della missione, hanno conosciuto il valore,

tutti coloro che hanno avuto anche un minimo contatto e che hanno dato un apporto alla nostra missione italiana devono essere accolti in Italia, senza se e senza ma. Non sono immigrati di seconda categoria, ma persone che vogliono continuare a stare vicino a noi.

in questi anni, di andare maggiormente fino in fondo, di svolgere quel ruolo di pace, ma con mezzi ancora maggiori, per consentire che oggi l'Afghanistan non corresse il rischio, che corre, di ritornare a com'era vent'anni prima. Non lo so quello che succederà. So che oggi...

e da lì parte la missione: com'è stato ricordato, per la prima volta si utilizza l'articolo 5 del trattato della NATO, con uno Stato alleato che viene attaccato, e parte, con grandissima emozione e anche preoccupazione, una coalizione internazionale. Nasce dunque la missione Enduring freedom, che gli Stati Uniti hanno voluto inizialmente comandata da una *coalition of the willing*,

il collega La Russa, anche i nostri militari hanno combattuto, perché è stato un momento di grandissimo contrasto fra le forze internazionali e il terrorismo. C'è un elemento che ha contraddistinto il contingente italiano dall'inizio (lo ricordo nelle parole che mi disse il generale Del Vecchio, che è stato anche nostro collega e comandante della missione ISAF): in una delle primissime occasioni in cui l'ho incontrato, nel suo ruolo ancora di militare, diceva che era fondamentale, per combattere il terrorismo, avere la popolazione afghana dalla nostra parte.

L'odio nei nostri confronti non ci aiuta a conquistare la popolazione alla lotta al terrorismo. Questa è sempre stata la prima preoccupazione delle nostre Forze armate. Il ministro Guerini ha raccontato quante scuole, ospedali e pozzi sono stati costruiti, non perché le nostre Forze armate fanno cose

la situazione era oggettivamente drammatica dal punto di vista della diffusione del terrorismo e quindi si può capire anche quel tipo di scelta, ma su come si utilizzano i *boots on the ground* gli italiani hanno sempre qualcosa da insegnare al mondo. C'è un altro elemento che vorrei ricordare a quest'Aula. Nel momento in cui la coalizione internazionale arriva in Afghanistan e cominciano le prime vittorie sui talebani, si apre un processo democratico, ci sono le elezioni del 2004 e si apre una grande fiducia nell'opinione pubblica afghana. Le donne vanno a votare, tutti escono con il dito sporco di inchiostro per dimostrare che hanno votato, c'è stata una grandissima partecipazione, nella legge elettorale si decide che il 25 per cento degli eletti devono essere donne; una grande apertura di fiducia. Ma poi quei governi, a volte per incapacità o perché non si mettevano d'accordo, spesso anche per corruzione, non hanno corrisposto alle aspettative della popolazione afghana e piano piano la fiducia che la democrazia portasse davvero un cambiamento è venuta meno; e quindi, ad esempio, la partecipazione alle elezioni è scemata. La seconda considerazione che voglio fare (la prima è come si interviene come coalizione internazionale) è allora la per liberare dal terrorismo e costruire dei percorsi democratici diventa fondamentale non solo l'intervento delle forze militari, ma come si aiuta questo Stato a costruirsi davvero e a dare le risposte, in infrastrutture e in economia. Altrimenti rimane un'iniziativa

si è deciso di diminuire le truppe della coalizione internazionale. Nel frattempo, però, i signori della guerra continuavano a esistere, il PIL afghano continuava a essere per il 20-30 per cento collegato alla coltivazione del papavero da oppio del papavero da oppio e i signori della guerra di questo si alimentavano. Nella difficoltà dell'Afghanistan, anche questo è un elemento che si è cercato di contrastare, ma è stato difficilissimo. Alla nostra cooperazione era venuto in mente di sostituire la coltivazione del papavero da oppio con lo zafferano, perché comunque è un elemento di grande pregio. Ma, in una situazione così complicata, i signori della guerra andavano a distruggere le coltivazioni di zafferano; si è trattato quindi di un tentativo nobile, che però ha incontrato tutta una serie di difficoltà. Abbiamo fatto anche molti progetti di cooperazione, per esempio con le cooperative di lavoro femminili, perché le donne sono state - come è stato ricordato da molti - le più colpite dal regime talebano. Nelle città è stato più facile, ma l'Afghanistan è in gran parte composto da zone rurali. C'era solo una grande strada che lo univa e moltissimi villaggi non erano neppure raggiungibili. Quando Emma Bonino era Quando Emma Bonino era inviata europea, ci eravamo incontrati e lei stava seguendo le elezioni. Ricordo un episodio, che voglio citare anche qui. Una giovane donna afghana decide di candidarsi alle elezioni: raccoglie i soldi e le firme necessarie e poi si mette in viaggio con il fratello, perché

complicazione del processo democratico rispetto alla situazione dell'Afghanistan. Mi avvio alla conclusione. Grande ruolo dei nostri militari grande riconoscimento della loro capacità di intervenire con attenzione verso la popolazione, che non vuol dire non fare il proprio mestiere di militari, ma vuol dire avere quelle alleanze che servono a farlo meglio.

Per mia fortuna, quando avevo la responsabilità del Ministero, non ho dovuto ricevere soldati morti in missione. Ma ricordo, perché ho partecipato a tutti i funerali, l'incontro con queste famiglie straziate dal dolore; è un dolore incredibile, che non

che ricorda tutte queste nostre vittime. *(Applausi)*. Credo che sarebbe giusto per ricordare il loro sacrificio e il loro straordinario eroismo nell'intervenire in quella situazione.

nella Conferenza dei Capigruppo. Siccome, però, c'è stato un lungo periodo in cui lasciavo sempre finire a tutti

motivo per cui siamo arrivati, d'accordo con tutti i Gruppi, alla determinazione che ci si debba tarare sul tempo che è stato prefissato perché poi si spegne automaticamente il microfono.

a tenere conto dei tempi stabiliti e a tarare il vostro discorso sui tempi per non dar luogo alle polemiche che voi stessi avete generato. A me dispiace francamente ogni volta vedere un certo disappunto quando non si termina il proprio ragionamento. Presidente, ringrazio il Ministro per la sua informativa che ci ha dato molti elementi e molte

perché credo che ci troviamo di fronte a un quadro, come molti interventi hanno sottolineato e come lei stesso, Ministro, ha fatto, che lasciamo in Afghanistan pieno di incognite.

Ovviamente lei sa, dal momento che in quest'Aula conosciamo le storie di tutti, che io avevo molti dubbi su quella missione; dubbi su cosa? Sull'idea che si potesse, come poi è avvenuto anche per l'Iraq, esportare la democrazia in questo modo. Devo dire che dopo venti anni,

Il lavoro che le Forze armate italiane hanno fatto, non solo in Afghanistan ma anche da altre parti, si è sempre contraddistinto perché noi siamo stati vicini alla popolazione civile, abbiamo fatto delle operazioni molto importanti proprio per aiutare la popolazione civile e per favorire i diritti. Ecco penso che questa debba essere la nostra

iniziative e continuare a lavorare perché faticosamente i diritti delle donne, i diritti umani...

nell'arco di venti anni, con un impegno importante, con tante donne e uomini che si sono misurati sul campo. Siamo stati apprezzati da tutti e, quindi, oltre ad aiutare quella popolazione, certamente tale missione è stata un'occasione per dimostrare, come del resto è avvenuto in altre missioni internazionali, che le nostre Forze armate rispondono al momento della chiamata, hanno saputo modernizzarsi e acquisire una capacità di intervento ampia. Tanto è vero il Gruppo di Forza Italia ha sempre votato a favore delle missioni militari internazionali di pace sia quando è stato in maggioranza, sia quando è stato all'opposizione e talvolta, quando il voto poteva servire a salvare un Governo che contrastavamo su altri campi, non abbiamo esitato a dare il nostro voto, che era un voto al ruolo internazionale dell'Italia e a sostegno delle nostre Forze armate. Lo abbiamo sempre

quindi è stato una risposta a un attacco immaginabile. Non avremmo immaginato di trovarci con delle mascherine sul volto nelle nostre città a causa di una pandemia planetaria, meno ancora avremmo immaginato che degli aerei si infilassero dentro i grattacieli di New York. Il millennio ci riserva sorprese tragiche e difficili, che vanno fronteggiate in modo diverso. diverso. Noi abbiamo fatto quella missione e la NATO è cambiata un po', non nella sua natura: lei ha citato anche l'articolo in base al quale la NATO ha deciso di intervenire, però non l'aveva fatto prima, quindi è stata una vicenda eccezionale.

il Governo Ghani ha dovuto cambiare il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa in questi giorni; c'è una situazione di difficoltà. Lei ha fatto riferimento ai droni, ai Paesi confinanti nei quali faremo attività addestrative, ma noi per la verità non sappiamo cosa accadrà.

però quando se ne andarono tutti, il Vietnam del Nord conquistò tutto e il disegno di Ho Chi Minh si realizzò. Io non vorrei che in Afghanistan si ritornasse a questo e che quindi si vanificasse il sacrificio umano, di vite ed economico della comunità internazionale. I dati della crescita delle

io ero tra quelli che inneggiavano ai *mujaheddin,* che allora erano chiamati così, non li chiamavamo talebani, il termine non era entrato in vigore. I *mujaheddin* erano i campioni della libertà che si battevano contro l'esercito.

quel Paese a una stagione di nuovo oscurantismo? Noi siamo molto preoccupati di quello che può accadere e lo dico affinché rimanga nel Resoconto a futura memoria; non vorrei che fra qualche anno alla fine i nipoti di Bin Laden o i nipoti dei *mujaheddin* (che allora vedevamo in un'altra maniera),

drammatica, arriva anche alle moschee clandestine che ci possono essere nelle nostre città: è una filiera. È vero che la vicenda che fa tanto scuotere le coscienze in questi giorni ha origine dal Pakistan, ma sono culture confinanti e vicine. Mi riferisco, a proposito dei diritti delle donne, a quello di cui discutiamo in questi giorni in Italia, al caso di Saman, a situazioni che arrivano in casa nostra. Noi non dobbiamo imporre niente a nessuno, ma i valori della democrazia, della convivenza, dei diritti delle persone, a qualsiasi sesso e genere appartengano, sono un baluardo delle democrazie occidentali. Per questo, in quel 2001, andammo in Afghanistan e altrove: per affermare la vittoria della democrazia e della libertà sull'oscurantismo fondamentalista. Per questo 53 italiani sono morti: per affermare questi diritti. *(Applausi)*! La questione non si è chiusa. chiusa. Qual è la verità? Vorrei dire anche un'altra cosa sul piano parlamentare. Noi abbiamo votato decine di volte le missioni internazionali, come ho ricordato all'avvio del mio intervento; abbiamo varato una legge per limitare il numero delle votazioni: si fa una programmazione annuale, annuale, abbiamo approvato anche una legge quadro, posto che le missioni internazionali non sono più un fatto episodico, ma un fatto ordinario del nostro Paese. Ringrazio, a nome del nostro Gruppo ma credo sia un sentimento condiviso, tutti i nostri militari, donne e uomini impegnati in tutti i contesti internazionali con grande valore e grande abnegazione.

questa volta non c'è stato un dibattito parlamentare sulla questione del ritiro dall'Afghanistan. Si vota per la missione, ma forse ci vuole un dibattito con un voto anche sulla fine della missione. La verità è che gli Stati Uniti hanno assunto una decisione

il Parlamento ha preso atto di questa decisione, che si rifletterà sugli equilibri di pace internazionali, sulla ripresa del fondamentalismo, sulle ripercussioni nei Paesi occidentali e nelle nostre città della malapianta del fondamentalismo,

su un lungomare o da qualche altra parte? È un tema delicato, lo so, però c'è una schedatura internazionale di molte di queste persone. È vero che oggi la predicazione può raggiungere uno che è davanti al *computer*, diventa un invasato, esce di casa e sgozza con un coltello una persona. Però ci sono alcuni soggetti che sono conosciuti e individuati. Dovremmo anche bilanciare: c'è un disimpegno sul territorio, quindi la comunità internazionale dovrebbe difendersi di più all'interno dei propri confini. La questione è lunga e complessa, il mio microfono lampeggia e la Presidente ci ricorda giustamente il rispetto dei tempi. Quindi, sottolineo l'omaggio alle Forze armate, l'apprezzamento alle missioni e ai militari che tornano, il rammarico per l'assenza di un dibattito parlamentare - ma è una critica generale al sistema, non un'accusa al Ministro - sul disimpegno, visto che noi votiamo frequentemente il rinnovo dell'impegno. È un monito alla comunità internazionale: non andiamo via perché abbiamo vinto, ma andiamo via perché andiamo via, e Dio voglia che non abbiano vinto gli altri.

innanzitutto un ringraziamento al nostro Ministro per l'informativa e per il lavoro che sta portando avanti. Mi unisco a lei nel commemorare i nostri caduti e nel celebrare il valore delle nostre Forze armate. Ho sentito una frase del presidente Casini: la politica estera del nostro Paese è portata avanti dalle nostre Forze armate; è giusto che sia così: la grande strategia di un Paese è fatta dalla politica estera e dalla politica della difesa. Parlo con te e ti mostro i muscoli; sono forte e disposto al dialogo: questa dovrebbe essere la realtà, ma molto spesso forse non parliamo nella maniera corretta; cerchiamo almeno di costruire un corpo muscoloso. Su questo ho fiducia nel nostro Ministro. Sono passati vent'anni e tutti hanno ricordato l'11 settembre. Io ricordo il marzo 2001: vi ricordate i Buddha di Bamiyan? Due grandi statue, patrimonio dell'UNESCO, che i talebani hanno voluto distruggere con l'artiglieria antiaerea e la dinamite; ci hanno messo settimane, ma sono riusciti a polverizzarli. India e Giappone, separatamente, hanno offerto del denaro

2001: un Paese in cui alle donne non era permesso vivere come esseri umani; giustamente molti hanno posto l'accento sul fatto che non potevano imparare a leggere e scrivere e non potevano esprimere se stesse come individui e come essere umani. La musica era proibita. Definire l'Afghanistan al livello del Medioevo è offensivo nei confronti dell'Europa del Medioevo, che non era così, pur avendo qualche problema di diritti umani, secondo il contemporaneo vivere.

mezzi antincendio per l'aeroporto di Herat, sostegno all'agricoltura, medicinali, cibo e così via. Abbiamo fornito sia la canna da pesca che il pesce, secondo un vecchio adagio, nel senso che abbiamo cercato di sostenere cioè i bisogni immediati e di fornire le strutture e i mezzi affinché quei bisogni venissero soddisfatti autonomamente dal popolo.

e gli Hazara, che tutti dimenticano, l'unica etnia sciita dell'Afghanistan, contro la quale tutte le altre etnie afgane provano odio, nient'altro che odio. L'Afghanistan è difficile da pacificare: quello che è stato fatto fino ad oggi, in questi vent'anni, è sicuramente un miglioramento. La soluzione non ce l'aveva in tasca nessuno. Del resto, voglio ricordare che quando la NATO, in particolare il Consiglio del Nord Atlantico, nel 2001 approvò l'intervento *ex* articolo 5, quindi la missione, non diede delle direttive strategiche, limitandosi ad un: armiamoci, partiamo e ogni Paese decide la linea da tenere. Non era la premessa ideale per vincere una guerra perché, se io combatto, lo faccio per un obiettivo, ma se non ho l'obiettivo...

con la decisione americana di inviare in maniera permanente una flotta, al fine di contenere la Cina, che rivendica che rivendica l'intero Mar Cinese meridionale come acque territoriali, in spregio alle convenzioni internazionali del XX e XXI secolo, nonché in spregio al principio banale di sovranità di Paesi come il Vietnam e le Filippine, che sono assolutamente sovrani.

ma siamo a livello di dover fare contenimento rispetto a una potenza revisionista, cioè che non accetta l'ordine mondiale esistente, e che può essere revisionista con ogni mezzo. *(Applausi)*. Di certo adesso vi starete chiedendo che cosa c'entrano i talebani in Afghanistan con la Cina. Benissimo, guardate la carta geografica

ci sono rapporti delle autorità di pubblica sicurezza cinese che parlano di attività talebane che stanno addestrando gli uiguri a difendersi dall'oppressione cinese.

nel Pakistan centrale, un'autobomba con un *kamikaze*. L'obiettivo dei talebani pakistani che rivendicarono questo attentato era l'ambasciatore cinese.

della Cina. La missione in Afghanistan è troppo costosa per la maggior parte dei Paesi occidentali (non tanto perché non possiamo, ma forse perché le nostre opinioni pubbliche non vogliono)

ringrazio anzitutto per la sua relazione. Il MoVimento 5 Stelle accoglie con grande gioia la decisione di ritirare finalmente le nostre truppe dall'Afghanistan, perché questa è stata la prima richiesta politica che il nostro movimento fece quando entrò in Parlamento nel 2013, con la sua prima mozione. una richiesta che abbiamo reiterato negli anni e che aveva già portato a una sensibile riduzione del nostro contingente militare. Questa storica decisione concordata con i nostri alleati mette fine a una delle guerre più lunghe e assurde della storia recente: una guerra punitiva, decisa dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 contro il Paese sbagliato (le responsabilità andavano individuate in altri Paesi, come Pakistan e Arabia Saudita) e contro un regime - l'Emirato islamico dei talebani - che di fatto ha resistito a vent'anni di occupazione e che, dopo il ritiro, si appresta a tornare al potere.

creando milioni di nuovi profughi e sostenendo un regime di criminali di guerra, integralisti e narcotrafficanti che hanno inondato di eroina il pianeta e lo stesso Afghanistan, con conseguenze sociali e sanitarie disastrose, che si sommano a povertà estrema e a una qualità della vita che è migliorata solo per una ristrettissima minoranza urbana (quella che si è arricchita grazie all'indotto dell'occupazione militare e umanitaria). Altro che esportazione della democrazia, la quale si impone non certo con la forza delle bombe, ma con la forza del pensiero e della cultura. una guerra sanguinosa, costata un numero enorme di morti da parte afgana: almeno 50.000 civili, secondo le stime più conservative, 65.000 membri delle forze di sicurezza locali e almeno altrettanti combattenti della resistenza talebana. Molti, troppi sono stati i morti anche da parte occidentale: oltre 3.500 soldati della NATO e almeno 4.000 *contractor*. Anche il nostro Paese ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite: 53 soldati caduti e oltre 700 feriti e mutilati, a cui va il nostro sentito e sincero ricordo. Oggi forse ci sono state troppe lacrime di coccodrillo; la realtà è che i militari hanno subito e pagato le scelte della politica, di cui ci si deve assumere la responsabilità. Ministro, colgo l'occasione per chiederle un suo personale impegno affinché la Difesa faccia piena luce sulla vicenda del caporal maggiore scelto David Tobini, parà romano morto a ventotto anni durante una battaglia contro i talebani in una trincea sul fronte di Bala Murghab, il 25 luglio del 2011, probabilmente vittima di fuoco amico. È recentemente emerso che il giovane pochi giorni prima aveva scritto una lettera alla madre, che dopo la sua morte venne presa in custodia delle autorità militari e mai consegnata alla madre di David. Perché questo? Signor Ministro, lo Stato ha onorato il sacrificio del soldato Tobini insignendolo *post mortem* di medaglie al valore e alla memoria; onoriamolo facendo giustizia. De Andrè, nella sua «Ballata dell'eroe», la splendida canzone contro la guerra, giustamente sentenziava: «Troppo lontano si spinse a cercare la verità. Ora che è morto la patria si gloria d'un altro eroe alla memoria. Ma lei che lo amava aspettava il ritorno d'un soldato vivo. D'un eroe morto che ne farà, se accanto nel letto le è rimasta la gloria d'una medaglia alla memoria»? Se i costi umani di questa guerra sono stati pesantissimi, lo sono stati anche quelli finanziari: oltre 2.000 miliardi di dollari sono stati spesi solo dagli Stati Uniti, più tutti quelli spesi dagli Alleati; dai 25 miliardi di euro del Regno Unito agli oltre 8,5 miliardi di euro pagati dai contribuenti italiani. Se si fosse spesa una frazione minima di questi capitali non per distruggere l'Afghanistan a suon di bombe, ma per ricostruirlo e aiutarlo, oggi quel Paese sarebbe la Svizzera dell'Asia centrale. Per non gettare al vento questo sacrificio di vite e risorse e per evitare che l'Afghanistan sprofondi in una nuova guerra civile, dopo il ritiro non dobbiamo assolutamente abbandonare il popolo afgano. L'Italia rimanga in prima linea per lavorare alla riconciliazione nazionale con i talebani, alla ricostruzione del Paese e a una rafforzata cooperazione civile allo sviluppo e per la tutela dei diritti umani. Facciamo oggi quello che avremmo dovuto fare vent'anni fa: investiamo risorse non più per la guerra, ma per la pace. A questo proposito, valutiamo bene l'opportunità di proseguire l'ingente sostegno finanziario italiano all'esercito afgano (circa 120 milioni di euro all'anno), che non farebbe altro che prolungare una sanguinosa guerra civile, una guerra per procura dall'esito già segnato. Dall'inizio del ritiro delle truppe NATO le forze talebane, che già negli anni passati avevano ripreso il controllo di gran parte dell'Afghanistan, stanno riconquistando distretti a un ritmo esponenziale e si preparano a entrare a Kabul. un'ipotesi così concreta che il Pentagono per scongiurarla sta già ipotizzando un nuovo intervento. Signor Ministro, non possiamo ripetere ancora gli stessi errori. Indiani, greci, arabi, mongoli, britannici, sovietici e americani: nessuno è mai riuscito a conquistare quel Paese, che non a caso si è guadagnato la fama di "cimitero degli imperi". Basta guerre. Lavoriamo piuttosto per favorire la riconciliazione nazionale, il disarmo dei ribelli e la loro reintegrazione, l'inclusione dei *pashtun*, che sono la maggioranza etnica del Paese, nel governo di un nuovo Afghanistan federale. Questa deve essere la nuova missione italiana e occidentale in Afghanistan, una vera missione di pace che il MoVimento 5 Stelle sosterrà con piena convinzione.

ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno.

oggetto del *question time* e cioè la questione riguardante i pagamenti della pubblica amministrazione ai fornitori di beni e servizi. Seppure in questo anno la situazione è oggettivamente migliorata, secondo i dati forniti proprio dal suo Ministero, credo ci siano ancora forti criticità, visto che nel 2020 sono stati 5.687 gli enti pubblici che hanno pagato in ritardo i propri fornitori, in 2.138 casi la pubblica amministrazione ha superato di un mese i limiti fissati dalla legge e in 229 casi ha superato di cento giorni le scadenze e il confronto è effettuato rispetto ai trenta giorni, sessanta per la sanità, previsti dalla normativa europea. Ad essere in ritardo nei pagamenti è ancora il 31,7 per cento delle pubbliche amministrazioni censite. Si spiega così l'aumento dei debiti commerciali pubblici, da 48,9 miliardi di euro, nel 2019, ai 51,9 dello scorso anno. Il Ministero dell'interno nel 2020 ha visto scadere oltre 390.000 fatture, per un valore complessivo pari a 2,43 miliardi di euro e ha pagato l'81,7 per cento con un ritardo medio di diciotto il Ministero della giustizia ha liquidato il 75,4 per cento delle fatture con un'attesa media di 17 giorni rispetto alle tempistiche di legge; nonostante l'Italia abbia recepito la normativa europea, è di tutta evidenza come risultino ancora difficoltà nella sua applicazione completa, e l'anno scorso l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per tali motivi, rischiando pertanto sanzioni se non riuscirà a limitare questi ritardi, capaci di ledere il diritto delle imprese al pagamento in tempi certi; il commissario straordinario per l'emergenza COVID, che ha fatto acquisti per 2,03 miliardi di euro, ha evaso pagamenti unicamente per una cifra pari a circa 1,15 miliardi (il 56,6 per cento) con tempi di attesa non performanti, pari in media a 15 giorni di ritardo; rilevato che il rispetto delle scadenze è un fattore di cruciale di cruciale importanza per il buon funzionamento dell'economia nazionale e rientra nel rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali, su cui la Commissione europea effettua un puntuale e rigoroso controllo, le chiedo, signor Ministro, di sapere quali urgenti iniziative il Ministero intenda adottare, al fine di sopperire ai ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione, a maggior ragione oggi, in cui dobbiamo organizzare anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Signor Presidente, la questione dei ritardi nei tempi di pagamento della pubblica amministrazione è da anni fonte di preoccupazione, in primo luogo per i problemi di liquidità e di svantaggio competitivo delle imprese italiane. L'obiettivo era ed è quello di assicurare il pieno rispetto della direttiva europea. Come ricordato dagli interroganti, da anni vi è un costante progresso nei tempi medi di pagamento. Il miglioramento è stato generalizzato, ma persistono alcune criticità, con alcune amministrazioni dello Stato e alcuni enti locali che registrano ritardi significativamente superiori al dato medio nazionale. Nel corso degli ultimi due anni sono state avviate diverse attività per migliorare la gestione dei pagamenti commerciali da parte delle strutture amministrative dei Ministeri e degli enti locali e per affrontare le aree di ritardo. Sono state convocate riunioni tra il MEF e i rappresentanti dei Dicasteri con maggiori criticità; questa azione ha consentito di ridurre il loro ritardo medio ponderato a dieci giorni nel 2020, sei in meno rispetto al 2019. D'intesa con l'ANCI, nel corso dello scorso anno sono stati organizzati *webinar* dedicati agli enti locali e incontri bilaterali con alcuni dei maggiori Comuni. Il ritardo medio ponderato nel corso del 2020 è sceso a circa quattordici giorni, tre in meno rispetto al 2019. Tali attività sono state intensificate nel 2021. Più recentemente, il decreto sostegni *bis* ha incrementato di un miliardo il fondo per assicurare la liquidità degli enti territoriali per i pagamenti dei debiti commerciali maturati a fine 2020. Da quest'anno sono entrate in vigore le misure finalizzate a incentivare il rispetto dei termini di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni non statali, che prevedono, in caso di inadempimenti, interventi correttivi proporzionali all'entità del ritardo. Circa la gestione commissariale per l'emergenza, il decreto-legge n. 73 di quest'anno ha autorizzato la spesa di un miliardo e 650 milioni per il pagamento di fatture pregresse, da trasferire al commissario previa presentazione da parte dello stesso di un rendiconto amministrativo susseguente al passaggio di consegne con la precedente gestione commissariale. La nuova gestione commissariale per l'emergenza ha ricevuto dall'inizio dell'anno 8.640 fatture, per un importo totale di 1,4 miliardi, a fronte dei quali sono stati pagati ad oggi 921 milioni (i due terzi), con un ritardo medio di circa un giorno. Il Governo è impegnato per proseguire nel miglioramento dei tempi di pagamento, con interventi sempre più mirati e selettivi per l'individuazione e la risoluzione delle specifiche criticità riscontrate. Continueremo inoltre ad assicurare la massima trasparenza sulle pagine dedicate del sito del MEF e a potenziare l'attività di monitoraggio e di supporto tecnico all'amministrazione. PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il Presidente, mi dichiaro soddisfatto della risposta del Ministro, perché credo ci sia la consapevolezza della necessità di questo intervento da parte del Governo. intervento da parte del Governo. I ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione hanno infatti un fortissimo impatto sulla vita delle imprese, sull'occupazione e sull'economia reale. reale. Riuscire a essere efficienti, oltre a essere un biglietto da visita per un Paese che è efficiente in Europa e che non si presta a pagare penali dovute al mancato rispetto dei tempi dei pagamenti,

e la messa in sicurezza di migliaia di posti di lavoro credo sia un limite forte che non possiamo permetterci, a maggior ragione se dobbiamo attrezzare la nostra struttura e organizzare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede fortissimi investimenti; anche lì i pagamenti nei confronti delle imprese private dovranno avvenire nel rispetto dei tempi

speciali in alcune aree del Paese, in particolare nelle Regioni definite meno sviluppate e in quelle in transizione. Si tratta sostanzialmente di Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania; ci sono poi le tre Regioni in transizione. Rispetto a queste Regioni, noi oggi abbiamo otto zone economiche speciali che sono state insediate. Abbiamo anche determinato, con idonea attività normativa, l'individuazione di commissari straordinari, che diventano interlocutori univoci delle attività delle imprese e degli enti locali. Si è determinato anche un raddoppio delle coperture finanziarie per quanto riguarda la prima attivazione. C'è bisogno adesso di concepire la reale attivazione di queste straordinarie zone differenziate per quanto riguarda l'attività della pubblica amministrazione nei confronti dei progetti di vita delle imprese.

possiamo fare in modo che parta un progetto con particolare dedizione al Mezzogiorno d'Italia per fare sì che aumentino le convenienze fiscali di credito di imposta e di alleggerimento degli oneri tributari in relazione a quei progetti di vita di impresa che sono capaci di generare aumento occupazionale? Le imprese chiedono semplificazioni, contenute nelle norme riguardanti le ZES; chiedono forme pattizie per fare in modo che l'obiettivo della vita dell'impresa sia anche obiettivo della vita istituzionale.

Signor Presidente, con riferimento alla richiesta dei senatori interroganti è importante sottolineare, come peraltro richiamato nel testo dell'interrogazione, che le attività economiche esercitate nelle ZES godono del credito d'imposta potenziato e introdotto nel 2017 in relazione agli investimenti in beni strumentali e che tale agevolazione è stata ulteriormente rafforzata con il decreto-legge semplificazioni di qualche settimana fa attraverso l'incremento del limite massimo dei costi ammissibili per progetto e mediante l'estensione dell'ambito oggettivo all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti. Nel valutare un ulteriore potenziamento del credito d'imposta per investimenti vanno tenuti in considerazione i vincoli istituzionali di natura europea. Va, infatti, garantito il rispetto degli specifici limiti e condizioni previsti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato e, in particolare, dal regolamento generale di esenzione dall'obbligo di notifica. Sempre per il rispetto della normativa europea non risulta possibile introdurre agevolazioni in materia di IVA e accise. A riguardo, si deve considerare che con la legge di bilancio per il 2021 la riduzione al 50 per cento dell'imposta sul reddito è stata riconosciuta in regime *de minimis* ed è difficilmente ipotizzabile che vengono ammesse ulteriori agevolazioni nell'ambito nell'ambito di tale regime. Per sostenere al meglio lo sviluppo economico delle ZES è essenziale garantire la rapida e piena attuazione di tutti quegli interventi amministrativi volti a creare condizioni ambientali idonee incentivare l'attività di impresa, potenziando la capacità amministrativa e alleggerendo gli oneri burocratici. Inoltre, la dotazione infrastrutturale è fondamentale. Seguendo questo approccio, il Governo ha deciso di destinare una quota delle risorse del PNRR allo sviluppo delle infrastrutture su porti e retroporti collocati nell'ambito delle stesse. Inoltre, significative risorse del Piano complementare sono destinate ai porti del Sud, in favore dello sviluppo dell'intermodalità e dei collegamenti dell'ultimo miglio e, più in generale, della capacità e della resilienza dei sistemi portuali. Queste iniziative saranno fondamentali per la creazione e lo sviluppo delle condizioni di contesto per consentire alle imprese di stabilizzarsi all'interno delle ZES e per e per permettere il recupero della competitività anche nei confronti dei porti concorrenti del Nord Africa e del Mediterraneo orientale. Il processo di potenziamento infrastrutturale sarà, inoltre, facilitato dalle semplificazioni procedurali introdotte dal recente decreto-legge n. che interessano anche la *governance*, ad esempio in materia di concessioni di autorizzazioni amministrative. In conclusione, gli incentivi fiscali già previsti e di recente rafforzati, uniti alle risorse per infrastrutture delle ZES e dei porti e alle semplificazioni, potrebbero permettere di affrontare alcuni fondamentali nodi critici dello sviluppo per le ZES. Ciò ovviamente richiederà un attento monitoraggio, al fine di verificare l'efficacia delle misure introdotte sull'economia delle zone del Mezzogiorno e di mettere a punto eventuali correttivi agli interventi.

soprattutto perché conosco la dedizione che ci sta mettendo la struttura del suo Ministero nel supportare il lavoro anche di altro Ministero dedicato e, in particolare, quello della coesione. Voglio mettere in evidenza che c'è una zona differenziata economicamente che funziona alla perfezione in Italia, caratterizzata dalla straordinarietà di una Regione. Il Friuli-Venezia Giulia ha una zona differenziata economicamente, amministrata da una figura di primo piano della nostra pubblica amministrazione, che è Zeno D'Agostino. Noi dobbiamo assumere le esperienze riuscite come esperienze di riferimento per quanto riguarda ciò che deve essere messo in cammino; coordinamento, monitoraggio, fare in modo che ci sia convergenza tra tutte le competenze dei soggetti competenti riguardanti lo sviluppo: evitare che Anas guardi da una parte e Ferrovie dall'altra, il sistema degli enti locali da un'altra parte ancora, con il demanio dello Stato che magari si chiama fuori. il coordinamento, il monitoraggio e la precisazione degli obiettivi programmatici. La zona economica differenziata è nata per fare in modo che lo sviluppo esca dalla nominalità e diventi realtà.

Presidente, signor Ministro, il decreto-legge sostegni *bis*, approvato dal Governo il 25 maggio di quest'anno ha stanziato ingenti risorse a sostegno delle imprese, del lavoro e del nostro sistema sanitario. Ha riproposto in particolare la misura del contributo a fondo perduto a favore delle partite IVA, che più di altre categorie sono state colpite dalle misure di chiusura rese necessarie dall'espandersi dell'epidemia e per motivi sanitari. In questa norma è stata opportunamente prevista la possibilità di vedersi accreditare sullo stesso conto corrente bancario dove è stato accreditato il precedente contributo un nuovo indennizzo, senza necessità di presentare un'ulteriore istanza da parte dei titolari di partita IVA che ne avessero i requisiti. Nelle settimane scorse il Governo ha comunicato alla Camera dei deputati che i contributi sarebbero stati accreditati in data 16 giugno e, successivamente, il 22 giugno, ha riproposto tale annuncio e tale impegno in un comunicato stampa. Stiamo parlando di circa 5 miliardi, essenziali per molte attività che hanno subito danni economici molto ingenti, hanno necessità di ripartire, di agganciarsi alla ripresa che si sta prospettando grazie alla stagione delle riaperture. Chi ha sofferto la stagione delle chiusure forzate va aiutato subito. La Lega ha apprezzato l'azione del Governo e l'impostazione del cosiddetto decreto sostegni *bis*, ma i bonifici a favore di questi titolari di partite IVA sembrano non arrivare in tempi congrui. Gli aiuti non vanno solo stanziati, ma anche erogati rapidamente. Chiediamo quindi al Governo le cause di tali ritardi, ma soprattutto se siano state finalmente superate e se i fondi verranno effettivamente erogati con celerità. Chiediamo inoltre quali siano gli intendimenti del Governo volti ad accelerare l'emanazione dei decreti attuativi previsti per affrontare l'emergenza economica e sanitaria che ha colpito il nostro Paese. Ci risulta infatti che degli 801 previsti, 471 attendano ancora di essere approvati. Non basta in definitiva stanziare risorse, non basta approvare buone norme, è fondamentale agire rapidamente. Chiediamo al Governo una risposta alla nostra interrogazione; la chiediamo perché chi ha sofferto la crisi economica più di altri ha diritto a risposte chiare e concrete.

delle istanze da presentare per l'erogazione del contributo a fondo perduto a beneficio degli operatori economici colpiti dall'emergenza Covid. In favore di questa stessa platea di beneficiari il decreto sostegni *bis* ha previsto l'erogazione automatica, senza la necessità di un'ulteriore istanza, di un contributo di ammontare uguale al precedente. Con riferimento a quest'ultimo contributo, preciso che, sebbene la norma non preveda un termine per l'erogazione del pagamento, tenendo conto degli elementi tecnici ed operativi dell'esperienza degli ultimi mesi, il 7 giugno, in sede di audizione sul decreto io stesso ho indicato nel 16 giugno la data in cui presumibilmente sarebbero partiti i pagamenti. Da successiva interlocuzione degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze con quelli della Commissione è emersa la necessità da parte di questi ultimi di approfondimenti sugli strumenti di monitoraggio approntati dai Paesi membri per il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19, il cosiddetto *temporary framework*. Non appena concluse tali verifiche, il Ministero dell'economia e l'Agenzia delle entrate hanno immediatamente attivato le procedure di pagamento che tecnicamente erano già state predisposte, dandone notizia attraverso la pubblicazione di un comunicato stampa il 22 giugno. Sono state già disposti 1.770.000 bonifici, con un controvalore di oltre 5 miliardi, cui si aggiungono altri 38.000 soggetti che si vedono riconoscere, sempre in maniera automatica, un credito d'imposta per complessivi 166 milioni. 166 milioni. Con riferimento al tema dell'attuazione dei provvedimenti emergenziali, siamo consapevoli che l'efficacia dell'azione di Governo dipende, oltre che dalla produzione di buone norme, anche dalla capacità di assicurare la tempestiva e piena operatività delle stesse. Su impulso della Presidenza del Consiglio le amministrazioni statali si sono dotate di una rete di monitoraggio e attuazione che sta intensificando gli sforzi nell'approvazione dei decreti attuativi e contestualmente sta operando una ricognizione sulle disposizioni normative risalenti nel tempo, di cui ad oggi non risulta ancora emanato il provvedimento attuativo previsto. Il MEF è investito di un numero di provvedimenti molto rilevante, considerato che il Ministero, oltre che essere proponente per i provvedimenti di propria competenza, è anche concertante o è chiamato ad esprimere pareri sulla maggior parte dei provvedimenti di competenza delle altre amministrazioni. Stiamo pertanto cercando di imprimere un'accelerazione ai ritmi con cui l'amministrazione sta operando al recupero dello *stock* normativo. Stiamo agendo su diverse linee d'azione, potenziando i sistemi di monitoraggio, rafforzando le strutture preposte ai provvedimenti attuativi introducendo nuove soluzioni organizzative.

perché si è affermato che le difficoltà sono state superate, quindi ci auguriamo effettivamente che dagli annunci si passi ai fatti, alla contribuzione a favore di chi è stato penalizzato più di altri da questa crisi. Tuttavia, continueremo a vigilare e a sollecitare l'Esecutivo affinché le norme approvate trovino un riscontro celere ed effettivo: questo è il nostro compito. La crisi sanitaria ha sicuramente colpito tutti indistintamente, ogni categoria, ogni area del nostro Paese e ogni fascia sociale. È stata terribile e ci auguriamo che, grazie alla campagna di vaccinazione, possa presto terminare in via definitiva. La crisi economica, tuttavia, non ha colpito tutti allo stesso modo: è innegabile che i lavoratori autonomi e titolari di partita IVA sono stati colpiti più di altri. Alcune categorie di lavoratori dipendenti hanno ricevuto correttamente e fortunatamente il proprio stipendio ogni mese; altri non hanno potuto lavorare, le loro attività sono rimaste chiuse, non hanno guadagnato, ma hanno dovuto continuare a pagare quanto dovuto al fisco e ai propri creditori. creditori. Queste categorie vanno quindi aiutate subito e costantemente. La Lega ha accolto le loro legittime richieste e le loro istanze di sostegno e si aspetta che vengano risarcite adeguatamente, in quanto rappresentano di fatto il cuore della nostra economia. Sono piccole attività che danno lavoro, versano ingenti contributi al fisco e hanno contribuito in modo fondamentale alla crescita economica del nostro Paese. Vanno sostenute, vanno aiutate a sopravvivere e a riprendersi senza ulteriori ritardi.

Signor Presidente, signora Ministro, sabato scorso a Roma, presso la stazione Termini, uno straniero in evidente stato di agitazione ha dapprima terrorizzato i passanti, armato di un coltello di notevoli dimensioni, e poi, all'arrivo della Polizia, ha rifiutato di deporre l'arma e anzi si è rivolto in modo aggressivo e minaccioso nei confronti degli agenti stessi. A quel punto un agente, come è noto, ha dovuto rispondere all'aggressione sparando un colpo di arma da fuoco verso gli arti dell'aggressore ferendolo a una gamba e pertanto neutralizzandolo. Questo episodio, che non è certamente il primo di cui purtroppo le cronache si occupano, pone evidentemente due ordini di gravi problemi.

nei confronti delle quali difendersi risulta veramente molto difficile per i cittadini onesti e perbene. Oltre al tema della sicurezza nelle nostre città, ce n'è uno ancora più grave che riguarda le dotazioni dotazioni dei tutori dell'ordine e le Forze di polizia. In particolare, si è acceso in relazione a quest'episodio un dibattito sulla necessità di dotare al più presto di Taser e di altre forme di difesa personale (ad esempio, di videocamere di ripresa da porre sulle divise degli agenti, le cosiddette *body cam*), in modo che chi interviene possa farlo in piena sicurezza per sé e anche nei confronti dei terzi. Le chiedo dunque, signor Ministro, di sapere quali sono le iniziative per accelerare il più possibile le gare, che sappiamo essere in corso, per la dotazione dei Taser. Le chiedo altresì di sapere quali iniziative intende assumere per far sì che l'iscrizione dell'agente nel registro degli indagati, definito "atto dovuto", non possa però avere avere come conseguenza una ulteriore demotivazione degli agenti di polizia e delle Forze dell'ordine, che troppo spesso rischiano di passare dalla parte del torto dopo essersi sacrificati per difendere la sicurezza dei cittadini.

Signor Presidente, onorevoli senatori, gli onorevoli interroganti, con riferimento al recente caso avvenuto a Roma di un cittadino ghanese resosi responsabile di un episodio di violenza che ha richiesto l'uso di arma da fuoco da parte di un operatore della Polizia di Stato intervenuto per neutralizzarlo, chiedono di sapere tra l'altro lo stato delle procedure delle gare relative all'acquisizione dell'arma comune ad impulsi elettrici con cui dotare le Forze di polizia. Va precisato preliminarmente che il complesso procedimento di acquisizione di tale tipologia di arma, comunemente detta Taser, è stata preceduta da una fase sperimentale disposta per ovvi motivi precauzionali. In data 16 giugno 2020, con mio provvedimento e nelle more della definizione dell'*iter* di adozione del decreto di modifica del decreto del Presidente l'uso dell'arma comune a impulsi elettrici, il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è stato autorizzato ad impiegare per i compiti istituzionali la predetta arma a condizione che essa non ecceda le potenzialità offensive delle Forze di polizia. In fase di gara è stato tuttavia necessario effettuare ulteriori approfondimenti circa gli *standard* di sicurezza e tale esigenza ha determinato un rallentamento delle stesse procedure, che sono ora in procinto di concludersi. Il prossimo 29 giugno verranno a cessare gli effetti della clausola *stand still*, termine dilatorio tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto prevista dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici. Conseguentemente, diverrà possibile procedere all'aggiudicazione in favore dell'operatore economico

All'esito favorevole del collaudo la fornitura, pari a 4.482 armi a impulsi elettrici e relativi accessori, sarà distribuita sul territorio nazionale. Desidero precisare che, dopo la fase di sperimentazione, è stato anche predisposto il provvedimento di carattere normativo che consentirà l'introduzione a regime della tipologia di arma in questione tra quelle in dotazione alle Forze di polizia. Una volta ottenuta la distribuzione dell'arma, si procederà a fornire il sistema di videoripresa, *videocam*, *body cam* al personale formato, in quanto i due strumenti sono connessi l'uno all'altro. Riguardo alla segnalata esigenza di far sì che gli agenti di polizia impegnati nei servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni di piazza possano operare con la necessaria serenità, aggiungo che si sta valutando di dotarli di strumenti tecnologici adeguati.

parzialmente soddisfatto della sua risposta, in quanto le informazioni tecniche che lei oggi ci ha fornito, molte delle quali in realtà erano già di dominio pubblico, risolvono soltanto una parte del problema. La verità è che, ancora una volta, le lungaggini burocratiche poi vengono pagate da chi si trova in prima linea ad affrontare situazioni di questo genere. Personalmente, la ringrazio delle precisazioni che ci fanno ben sperare per il futuro, ma ormai il ritardo accumulato è quello che è, non lo possiamo certamente più recuperare. Signora Ministro, c'è un tema che avevo posto sul quale lei ha mantenuto un rigoroso silenzio ed è appunto come si possa evitare che l'iscrizione nel registro degli indagati degli agenti che fanno il loro dovere che fanno il loro dovere si trasformi in ulteriore demotivazione di chi deve affrontare fatti come questi che potrebbe poi sentirsi autorizzato, ad un certo punto, a girarsi dall'altra parte per evitare di correre il rischio di passare dalla parte della ragione alla parte del torto. del torto. Il paradosso è che in questo caso abbiamo un agente che ha fatto il suo dovere di servitore dello Stato e si trova a difendersi e a dover anticipare anche le spese legali per la sua difesa; dall'altra parte abbiamo l'aggressore, che improvvisamente diventa addirittura parte offesa e avrà le spese legali pagate dallo Stato due volte, una come imputato e una come parte civile nell'eventuale processo contro l'agente che ha fatto il suo dovere. Credo che siano paradossi ai quali dobbiamo porre finalmente rimedio.

Signora Ministro, il 18 e 19 giugno 2021, qualche giorno fa, io e la mia collaboratrice, l'avvocato Alessandra Ballerini, siamo stati in visita ispettiva all'*hotspot* di Lampedusa, dove tra l'altro - lo dico in via di premessa - ci sono state frapposte pesantissime ed indebite interferenze nell'espletamento del mandato parlamentare; nonostante la limpidezza del quadro normativo primario di riferimento. Ovviamente tali interferenze sono state immediatamente segnalate alla procura della Repubblica competente. Nella visita si sono evidenziate condizioni di invivibilità completa nell'*hotspot*, dove sono spesso costrette a vivere anche 2.000 persone, a fronte di una capienza di 228 posti. Queste persone - si ribadisce - sono trattenute nell'*hotspot* senza alcuna colpa. Centinaia di persone con 40 wc; uomini, donne e bambini giacciono all'aperto, all'aperto, anche di notte, nonostante lì il clima non sia affatto mite la notte. In questi giorni, oltre alle condizioni disumane, è emersa una completa abdicazione, signora Ministro, dello Stato che si manifesta in innumerevoli incertezze, approssimazioni, discrasie. In primo luogo, c'è una completa discrasia di opinione circa il regime cui sono sottoposte le persone che sono concentrate nell'*hotspot*. In particolare, non è dato capire se quelle persone possono lasciare liberamente il luogo di concentrazione in cui sono chiuse, oppure no. Infatti, i militari dell'esercito che sono al corpo di guardia, incaricati della sorveglianza degli ingressi, riferiscono che non si possa uscire. Le persone presenti nell'*hotspot* non hanno quindi libertà di movimento. Al contrario, alcuni elementi della Polizia hanno sostenuto che gli ospiti possono allontanarsi; altri sostengono il contrario. Insomma, si va a una vera e propria dematerializzazione dematerializzazione e confusione che volgono verso un'anarchia a trazione poliziesca. Non c'è un regolamento che possa fare da riferimento e criterio a queste cose. Non risulta, inoltre, alcun criterio predeterminato per la distribuzione delle persone a bordo delle costosissime, antieconomiche, inefficaci e inutili navi quarantena, oppure la destinazione verso altri luoghi di trattenimento o di concentrazione.

le situazioni di afflusso massimo di migranti. Sono strutture previste dal diritto eurounitario già da qualche anno. Gli *hotspot*, tuttavia, non rappresentano in alcun modo delle strutture detentive, cioè strutture nelle quali il migrante viene privato della sua libertà personale. A tale funzione corrispondono i centri di permanenza per i rimpatri Negli *hotspot,* tuttavia, vengono effettuate quelle operazioni di polizia (identificazione, fotosegnalamento e rilevazione delle impronte digitali per il loro inserimento nella banca dati Eurodac), come impone il regolamento dell'Unione europea, a protezione delle frontiere esterne, e di soccorso e *screening* sanitario che richiedono il trattenimento del migrante per un limitatissimo periodo di tempo, necessario all'espletamento delle predette funzioni. Come noto, l'*hotspot* di Lampedusa è periodicamente oggetto di sovraffollamento, che tuttavia viene efficacemente fronteggiato con un rapido decongestionamento delle situazioni eccedentarie, come ha potuto constatare lo stesso senatore De Falco. In effetti, il senatore De Falco ha fatto accesso all'*hotspot* di Lampedusa il giorno appena seguente alla sua richiesta, in quanto il giorno prima si era verificata una situazione di particolare sovraffollamento (in poche ore affrontata e risolta), che rendeva controindicato, anche per ragioni sanitarie, il richiesto accesso. Non corrisponde pertanto a realtà che il successivo trattamento del migrante risponda a criteri casuali, come sostengono gli interroganti. È vero, viceversa, che ciascun migrante, una volta effettuate le preliminari operazioni di polizia e *screening* sanitario, oggi anche in funzione Covid, riceve un trattamento adeguato alle sue condizioni e al suo *status,* anche e soprattutto con riguardo alle posizioni di vulnerabilità che concernono i nuclei familiari e i minori non accompagnati. Peraltro, l'attenzione verso i diritti umani e la preservazione della dignità dei migranti sono testimoniate non solo dal quotidiano sforzo degli operatori di polizia presso le strutture, ma anche dal forte coinvolgimento delle organizzazioni umanitarie. Esse operano in base a convenzioni con il Ministero dell'interno a tutela e sostegno del migrante e rispondono ai nomi di UNHCR, OIM, Save the children e Medici senza frontiere. frontiere. Analoghe condizioni di tutela del migrante vengono garantite anche a bordo delle navi dalla Croce Rossa proprio per assicurare l'assistenza sanitaria e l'apprestamento delle cure necessarie per i migranti ivi ospitati.

penale, ossia con una pesantissima interferenza. Io sono stato ammesso il giorno seguente. Io sono stato a Lampedusa il 18 e il 19 giugno, avendo già preavvertito in precedenza il prefetto

e le decisioni di coloro che decidono della libertà delle persone che sono lì trattenute. Quelle persone sono lì trattenute, signora Ministro: non c'è alcuna libertà di uscire ed entrare, nessuna. Tanto è vero che mi è stato impedito di entrare, quindi non diciamo cose inesatte. Le cose non vere vengono dette da lei, signora Ministro, e dall'amministrazione purtroppo. Voglio soltanto sapere cosa intende fare, in linea generale, per assicurare umanità in quel posto: 950 persone, ridotte a 450 (non a tre, signora Ministro), sono state per metà portate sulla nave Atlas e per metà sono rimaste lì, a vivere all'addiaccio, tra i topi. È questa la civiltà che noi vogliamo esportare, di cui ci vantiamo, signora Ministro? Lei su questo non ha risposto e non ho altro da aggiungere.

volti a limitare le partenze dalle coste africane e a intervenire da un punto di vista normativo, per quella che è la nostra competenza, per impedire alle organizzazioni non governative di agire in modo tale da facilitare l'attività dei trafficanti di persone, bloccando anche gli sbarchi.

queste persone si dedicano ad attività di carattere criminale, anche solo per sopravvivere, e vanno ad incrementare soprattutto lo spaccio, quindi il deterioramento complessivo delle nostre città.

non riferire non solo un allarme sociale, ma anche una chiarissima problematica di sicurezza, di tranquillità, sia per quello che riguarda le Forze dell'ordine, come le hanno ricordato alcuni colleghi prima, sia soprattutto per quello che riguarda i cittadini. La ringrazio e aspetto la risposta.

Signor Presidente, onorevoli senatori, gli onorevoli interroganti, con riferimento ai temi sollevati sottolineano innanzitutto la necessità di affrontare la questione migratoria ricorrendo alla stipula di accordi di partenariato con i Paesi di origine e di transito dei flussi. È noto come la linea a cui mi sono sempre attenuta, in ogni foro internazionale, a livello multilaterale e bilaterale, sia quella di sollecitare l'Unione europea a porre mano con urgenza ad accordi di partenariato strategico con i Paesi da cui si origina la pressione migratoria, a partire dalla Libia e dalla Tunisia. Peraltro, di tale sforzo è stato dato atto pienamente nelle proposte di risoluzione approvate ieri dal Parlamento, proprio in vista del Consiglio europeo, in programma oggi e domani a Bruxelles, sul quale ha riferito il presidente Draghi. di risoluzione si prefigura il superamento dell'ormai obsoleto quadro giuridico di Dublino, per porre il tema migratorio e della connessa solidarietà intraeuropea al centro dell'agenda dell'Europa. Altra priorità è il rafforzamento della cooperazione dell'Unione europea migrazioni (OIM), sul versante dei corridoi umanitari e su quello dei rimpatri volontari assistiti, quali strumenti utili per ridurre i flussi irregolari e contrastare il traffico di esseri umani nel Mediterraneo. Passando ora agli altri temi dell'interrogazione e in particolare alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, segnalo che con l'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, sono state implementate le misure di contrasto allo spaccio di stupefacenti all'interno e in prossimità prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico o di pubblici esercizi. A tutela soprattutto dei giovani è stato introdotto il divieto di accesso in esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento dei soggetti che abbiano riportato denunce o condanne per la vendita o cessione di stupefacenti. A completamento di tale misura è stato anche previsto che chi abbia precedenti per le stesse tipologie di reato non possa neanche stazionare nei predetti locali, proprio in forza del Daspo urbano. Rinviando per quanto attiene all'arresto obbligatorio in caso di spaccio agli ulteriori approfondimenti che potranno essere svolti con il competente Ministero della giustizia, aggiungo che recentemente ho licenziato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un decreto ministeriale che assegna ulteriori risorse ai Comuni, pari a 15 milioni di euro, per il triennio 2020-2022, proprio per potenziare le iniziative di prevenzione e contrasto alla diffusione delle droghe.

sono intimamente connessi con la coesione sociale, nel senso che non avere un occhio attento alla sicurezza, legata anche all'immigrazione, vuol dire dare la percezione di non essere altrettanto attenti alla parità della coesione sociale. Naturalmente siamo anche soddisfatti, perché abbiamo colto nelle sue parole e in quello che è stato detto anche ieri, che la l'attenzione del Consiglio europeo, su stimolo del Presidente del Consiglio, è concentrata sulle rotte migratorie, come parte integrante della politica dell'Unione

barche di morte. A questo proposito, è soprattutto importante che sia stato messo all'ordine del giorno questo tema, che dal giugno 2018 non era all'ordine del giorno del Consiglio europeo.

in collegamento a ciò, l'incertezza in cui si trovano 46 agenti della Polizia municipale, assunti con contratto a tempo determinato, in virtù delle risorse finanziarie che sono state assegnate al Comune di Messina con il Fondo nazionale

negli anni e che ha quindi determinato una grave carenza nell'organico. Una carenza che è stata resa ancora più evidente dalla maggiore rilevanza che hanno assunto i nuovi compiti di presidio e prevenzione sul territorio che gli agenti di Polizia municipale sono chiamati in tutta Italia a dover fronteggiare proprio nel caso dell'emergenza Covid, come supporto alla popolazione e come controllo del territorio. In altri termini, si è verificata di fatto un'espansione delle competenze delle Polizie municipali italiane, che rende oggi necessario riconsiderare le risorse stanziate in dotazione ai Comuni per gli organici, le strumentazioni e anche per un'adeguata formazione; organici, strumentazioni e formazione delle Polizie municipali appaiono evidentemente insufficienti, a fronte di una richiesta di incremento delle attività e dell'impegno della Polizia municipale, in considerazione delle complesse contingenze sociali connesse alla pandemia e al gravoso compito di far rispettare le disposizioni di contenimento relative alle norme Covid.

D'altra parte, è positivo il riscontro che si è avuto per le iniziative di sicurezza urbana finanziate con il fondo nazionale, che nel prossimo triennio assegnerà 65 milioni di euro a supporto dei Comuni che intendono potenziare il personale a tempo determinato delle polizie locali e la messa in sicurezza delle aree più problematiche delle nostre città. Quello che le chiedo è proprio se il Comune di Messina rischia a breve di vedersi privato di queste risorse e se quindi è possibile prorogare il contratto

Il Comune di Messina ha aderito al progetto «Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni», con risorse a valere sul Fondo per la sicurezza urbana 2018-2020, presentando, nel marzo 2019, un progetto per il potenziamento del Corpo di polizia municipale, che prevedeva, tra l'altro, l'assunzione a tempo determinato di 28 agenti di Polizia locale per l'anno 2019 e di 18 agenti per l'anno 2020. Il progetto è stato approvato in sede di Comitato ordine e sicurezza pubblica della prefettura di Messina e finanziato successivamente con decreto del Ministero dell'interno del 27 giugno 2019. Espletate le procedure concorsuali, il 13 agosto 2020 sono stati formalizzati 44 contratti individuali di lavoro a tempo pieno e determinato, con scadenza prevista al 13 agosto 2021. Poiché due vincitori avevano rinunciato all'incarico, è stato effettuato lo scorrimento della graduatoria e sono stati sottoscritti due ulteriori contratti di lavoro con scadenza 1° novembre 2021. L'assunzione di tale personale ha permesso il potenziamento delle attività di controllo e vigilanza sul territorio, con la partecipazione a operazioni interforze e un impiego importante anche nella gestione della crisi Covid-19. In relazione alla specifica richiesta formulata dall'onorevole interrogante, informo che le risorse del Fondo sicurezza urbana per il prossimo triennio 2021-2023 ammontano complessivamente a 15 milioni di euro per l'anno in corso e a 25 milioni di euro per l'anno 2022. Il decreto di ripartizione di tali stanziamenti, sottoposto preventivamente al vaglio della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato già concertato con il Ministro dell'economia e delle finanze e presto verrà licenziato definitivamente. In base ai criteri contenuti nel decreto, sarà attribuita al Comune

Con l'apporto di tali risorse il Comune potrà garantire la continuità dell'impiego degli operatori di Polizia locale anche eventualmente, ove ritenuto, implementandone il numero, come auspicato dall'onorevole interrogante.

Colgo l'occasione per ribadire e sottolineare l'impegno, la professionalità e la dedizione che il Corpo di polizia municipale del nostro Paese garantisce in sicurezza e controllo del territorio in questo difficile tempo di pandemia, pandemia, che ha messo un po' tutti su vari fronti a dura prova, proprio perché i nostri vigili urbani non sono solo coloro che gestiscono il traffico, la sosta e la viabilità, ma hanno tutta una serie di compiti e di deleghe importanti. In una visione più ampia, sono proprio la prima e più immediata interfaccia delle istituzioni con i cittadini. Sono coloro che vivono a stretto contatto con la comunità proprio nel quotidiano, raccogliendo suggerimenti,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, richiamo l'attenzione di questa Assemblea per segnalare una questione che mi sta particolarmente a cuore ed è oggetto anche di un'interrogazione che ho posto al Ministro della transizione ecologica, sottoscritta anche da molti colleghi. La questione riguarda la gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia, ma la sua rilevanza va ovviamente oltre i confini territoriali. Da sempre il tema rappresenta non solo in Sicilia un terreno di storica interferenza fra interessi privati e pubblica amministrazione. In questo momento storico di emergenza ambientale, sanitaria ed economica, la gestione dei rifiuti assume un rilievo politico e sociale più importante che mai. Non possiamo continuare a cercare soluzioni nel massiccio conferimento dei rifiuti in discariche private, né, come annunciato dal governo della Regione Siciliana, giocare con le leggi e con la salute e inaugurare una nuova stagione di costruzione di inceneritori, calata dall'alto, in barba alle direttive europee e a qualsivoglia processo decisionale e democratico. Se si intende costruire degli inceneritori al posto delle discariche, il governo regionale dovrebbe riscrivere daccapo il piano rifiuti, sottoporlo nuovamente al Parlamento e, soltanto dopo che tutto l'*iter* sarà concluso, presentare il bando per i termovalorizzatori. Come ebbe a dire l'allora ministro Costa, quando arriva un inceneritore o termovalorizzatore, il ciclo dei rifiuti è fallito. Raccolta differenziata, riuso e recupero sono i temi che dobbiamo portare avanti. È palese che la costruzione di nuovi inceneritori ostacola la prospettiva di un'economia circolare, principalmente caratterizzata dalla riduzione della produzione di rifiuti, progettati per poter essere correttamente differenziati, riciclati e recuperati.

Detto questo, ad un intervento di fine seduta deve seguire il lavoro o ci si illude che tutto si possa risolvere con la magia. Non si devono vendere illusioni, ma la prima cosa fondamentale consiste nel parlarne affrontando temi che nelle Aule parlamentari sono sempre stati avvolti da un velo di omertà. Si prestano entrambi a facili strumentalizzazioni e alimentano un dibattito più attento all'ideologia che ai diritti umani. Mi riferisco alla *cannabis* medica e all'eutanasia. Nel primo caso è bene chiarire che non stiamo parlando di stupefacenti, come qualcuno vorrebbe far credere, ma di una fondamentale sostanza terapeutica in grado di alleviare le sofferenze fisiche di centinaia di migliaia di pazienti. Inoltre si tratta anche di un settore ad altissimo potenziale per il nostro Paese. Come stimato dall'Istat, l'industria legata alla *cannabis* rappresenta lo 0,8 per Dal 2015 ad oggi la diffusione in commercio di *cannabis* medica non è andata di pari passo ad un costante aumento della domanda. Chiedo pertanto al Ministero della salute di attivarsi per garantire il diritto alla cura anche a tutti coloro che hanno bisogno di questa sostanza tramite l'individuazione di nuove fonti di approvvigionamento, preferendo l'apertura di nuovi siti produttivi nel nostro Paese, invece di puntare esclusivamente su un'importazione che comunque latita. Su un tema così importante è opportuno che si provveda ad attribuire una delega *ad hoc* sulle relative competenze senza menare il can per l'aia. Bisogna rendere concreta questa speranza. Speranza, batta un colpo. L'eutanasia invece è un argomento sul quale insiste un gravissimo vuoto normativo in grado di generare immenso dolore e sofferenza. La settimana scorsa sono rimasto profondamente colpito dalla storia di Daniela, una donna trentasettenne, paziente oncologica, che avrebbe voluto scegliere come morire, ma che non ha fatto in tempo a raggiungere una clinica in Svizzera. Sono tante le persone che prima di lei hanno dovuto sopportare e continuano a sopportare questo supplizio, una sofferenza disumana sia per la persona che per i familiari, ai quali va tutta la mia vicinanza. Entrambi questi temi rappresenterebbero delle conquiste di civiltà, nonostante alcune forze politiche preferiscano derubricarli a mere battaglie ideologiche. Visto che il nostro è uno Stato laico, mi chiedo quando troveremo nelle Aule parlamentari la forza per sgomberare il campo da polemiche ed ideologie e di occuparci finalmente di queste fondamentali tematiche in grado di alleviare o prevenire gravissime sofferenze. È umano uno Stato che non agisce davanti a queste immani sofferenze? È razionale trincerarsi dietro pregiudizi ideologici e culturali, arrivando finanche a sconfessare la scienza? Noi, come Movimento 5 Stelle, siamo pronti e lo siamo da tempo. da tempo. Martin Luther King ci ricordò che la libertà di ognuno di noi finisce là dove inizia quella degli altri. Porre ulteriori e irragionevoli limiti al diritto ad una cura e alla libertà di autodeterminazione non è una scelta politica, né ideologica,